L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

Quanto stiamo per approvare oggi in terza lettura - lo ripeto - è un provvedimento storico, doveroso e necessario per salvaguardare la coesione sociale di questo Paese. una misura che tanti altri Paesi europei hanno messo in atto da tempo e che viene proprio dall'esigenza di contrastare una situazione aggravatasi negli anni e precipitata durante la crisi economica internazionale che ha portato l'Italia a possedere il non invidiabile *record* del più alto tasso di incremento dei soggetti a rischio di esclusione sociale in Europa (un dato statistico che - di fatto - si tramuta in milioni di persone in povertà assoluta e in circa 10 milioni in povertà relativa). L'urgenza del provvedimento è confermata non solo dai dati ISTAT, ma anche e soprattutto dalle tantissime domande per accedere al reddito e alla pensione di cittadinanza che sono arrivate fino ad ora tramite Poste italiane e attraverso i Per la precisione, gli ultimi dati di Poste italiane ci parlano di oltre 220.000 domande. Le domande presentate tramite i CAF, invece, risultano essere oltre 500.000. Le richieste arrivano indistintamente da Nord a Sud. a Sud. Le città ove vi è un numero maggiore di richieste sono Milano, Torino, Roma, Napoli e Palermo. Si tratta di un provvedimento necessario anche - lo ribadisco - alla luce del pilastro europeo dei diritti sociali che all'articolo 14 statuisce: «Chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla reintegrazione nel mercato del lavoro». E appunto queste sono le finalità e la *ratio* del provvedimento, quindi perfettamente in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali. Si tratta di una misura di sostegno al reddito, ma non solo: una misura proattiva collegata all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo del cittadino, un grande investimento nei centri per l'impiego, nell'interoperabilità delle banche dati e nelle politiche attive del lavoro. Il reddito di cittadinanza costituisce dunque anche una grande innovazione delle politiche attive del lavoro e un importantissimo e necessario investimento nell'interoperabilità delle banche dati. Vengono, tra l'altro, istituite due piattaforme digitali propedeutiche al funzionamento il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e il Sistema informativo unitario dei servizi sociali per il coordinamento dei Comuni. Queste due piattaforme formeranno un grande portale unico per permettere la comunicazione e lo scambio di informazioni tra Comuni, Centri per l'impiego, Agenzie per il lavoro, ANPAL, Ministero del lavoro e INPS. Il lavoro parlamentare ha permesso di perfezionare un testo che era già efficace. Gli emendamenti approvati, sia al Senato che alla Camera, mirano a facilitare ancor di più l'accesso al reddito e alla pensione di cittadinanza. Inoltre, vanno incontro ad alcune categorie che più di altre in questi anni hanno subìto la crisi e le politiche di *austerity*, come i pensionati, le persone diversamente abili e i cosiddetti *working poor*, ossia persone che pur lavorando guadagnano talmente poco da non potersi permettere una vita dignitosa. Illustro brevemente alcuni degli interventi introdotti nel corso dell'esame in Senato. la definizione di offerta congrua fatta a un percettore di reddito di cittadinanza, che dovrà prevedere una retribuzione di importo uguale o superiore al 10 per cento in più di 780 euro.

restituire l'incentivo. È stata data la possibilità di esonero contributivo anche in caso di assunzione di persone in contratto di apprendistato. È stata disposta, in caso di dimissioni volontarie, la perdita del beneficio solo e unicamente da parte del dimissionario e non da parte di tutto il nucleo familiare. È stata prevista una modifica delle sanzioni ai CAF in caso di trasmissione infedele delle pratiche. Si è introdotta la previsione secondo cui i datori di lavoro che non sono in regola con la legge n. 68 del 1999 sul collocamento dei disabili, che determina le quote obbligatorie dedicate ai disabili, non potranno godere dell'incentivo. Infine, è stato previsto che le competenze acquisite dai beneficiari del reddito di cittadinanza saranno registrate sulle piattaforme. Si tratta quindi di uno storico delle competenze acquisite dal beneficiario del reddito in precedenti esperienze lavorative o percorsi di formazione e istruzione, che andrà inserito nelle suddette piattaforme completandone il profilo. Nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che il reddito di cittadinanza assuma la denominazione di pensione di cittadinanza oltre che nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a anche nell'ipotesi in cui uno o più componenti del nucleo possiedano il suddetto requisito anagrafico e convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. La Camera ha altresì elevato i limiti massimi del valore del patrimonio mobiliare con riferimento ai nuclei in cui siano presenti soggetti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza portando l'incremento da 5.000 a 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. È stato introdotto, inoltre, uno specifico innalzamento del parametro della scala di equivalenza (fino a 2,2) per l'ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti membri in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni relative ai redditi da pensione o da lavoro. È stato previsto l'incremento di cento unità della dotazione organica degli ispettori della Guardia di finanza e un incremento di 65 unità del contingente di personale per la tutela del lavoro dell'Arma dei carabinieri. Sono state introdotte diverse altre modifiche che riguardano le assunzioni da parte di Regioni, Province autonome, agenzie ed enti regionali: per la precisione, un aumento della dotazione organica fino a 3.000 unità con decorrenza dal 2020 e fino a 4.600 unità a decorrere dal 2021 del personale dei centri per l'impiego. Le quote inoltre includono la stabilizzazione delle unità di personale reclutate mediante procedure concorsuali bandite per le assunzioni con contratto a tempo determinato. Sempre con riferimento alle modifiche operate dalla Camera all'articolo 12, si ricorda che le risorse finanziarie in favore di ANPAL Servizi SpA, inerenti sia alla selezione di soggetti e alla conseguente stipulazione di contratti di collaborazione per concorrere all'organizzazione dell'avvio del reddito di cittadinanza, sia alla gestione delle spese, sono state previste in 90 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Si è precisato inoltre che la pensione di cittadinanza potrà essere ritirata alle Poste o in banca anche in contanti e non necessariamente essere caricata sulla carta del reddito. Numerose altre sono le proposte effettuate dai Gruppi di maggioranza e dai Gruppi di opposizione inserite all'interno del disegno di legge

Signor Presidente, in questa mia breve relazione mi limiterò a illustrare le modifiche e le integrazioni apportate alla Camera sugli articoli relativi a quota 100. L'articolo 14 è stato integrato con norme transitorie in materia di procedure concorsuali e di assunzioni del Ministero per i beni e le attività culturali al fine dichiarato di far fronte alle esigenze di sostituzione del personale, derivanti dall'ampliamento delle possibilità di pensionamento operato dal presente decreto e di assicurare la funzionalità degli uffici del Dicastero. In base a un analogo ordine di considerazioni, il comma 2 del successivo articolo 14-*bis* consente che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale procedano alle assunzioni, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengano in corso d'anno, fermo restando il rispetto della programmazione regionale e dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle Regioni di appartenenza. 14-*ter*, si ridefiniscono le modalità di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, con riferimento ai soggetti rientranti nelle categorie beneficiarie del cosiddetto collocamento obbligatorio. In merito alla possibilità di riscatto introdotta dai commi da 1 a 5 dell'articolo 20, per il triennio 2019-2021, con riferimento ad alcuni soggetti e fattispecie (riscatto relativo a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, né soggetti ad alcun obbligo contributivo), la Camera ha precisato che la domanda può concernere, fermi restando i suddetti presupposti, anche qualsiasi periodo temporale dei due anni in cui risultano accreditati, rispettivamente, il primo e l'ultimo contributo. Riguardo alla possibilità di applicazione di nuovi criteri di calcolo dell'onere di riscatto (sempre a fini pensionistici) dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo, possibilità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 20, la Camera ha soppresso il limite massimo anagrafico per il richiedente, limite posto dal testo originario del decreto-legge e pari a

Grazie Presidente. Sappiamo benissimo tutti che in questo passaggio al Senato il «decretone» dovrà essere solo ed esclusivamente convertito in legge così come ci è arrivato dalla Camera dei deputati, ovvero blindato, pena la decadenza del decreto stesso e la conseguente fine del Governo giallo-verde. La forzatura è stata evidente a tutti i livelli, a partire dalla scelta di procedere per decreto pur in assenza dei requisiti - lo ricordiamo - di straordinaria necessità e urgenza, al ricorso alla fiducia alla Camera dei deputati per limitare la discussione e l'emendabilità del provvedimento e riuscire così a rispettare la scadenza dettata dalle norme relative alla conversione in legge. forzatura persino nella comunicazione istituzionale effettuata attraverso la pubblicità in Rai. Dal 5 febbraio scorso si è venduto il reddito di cittadinanza come legge vigente mentre, in realtà, non è ancora legge, nemmeno in via provvisoria. Non solo si tratta di una comunicazione illegittima e non veritiera, a proposito di onestà e trasparenza, ma anche di una palese, inaccettabile svalutazione del ruolo del Parlamento. In sede di prima lettura, avevamo evidenziato come il testo presentasse carenze e ambiguità macroscopiche non solo formali ma anche sostanziali. In generale, le modifiche introdotte alla Camera dei deputati, numerose e complesse, tanto che gli articoli da 29 sono passati a 44 e le norme attuative da 24 a 38, impattano su un'operatività che è già stata avviata almeno dal 6 marzo scorso, generando delle criticità notevoli. In effetti, essendo stati modificati tra gli altri anche i requisiti e le condizioni per accedere al beneficio, sono state necessariamente introdotte delle norme transitorie all'articolo 13, comma 1-*bis*, ovvero per far salve le richieste presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, viene comunque riconosciuto il beneficio erogato per almeno sei mesi, pur in assenza di una eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti. Quindi, a tutte le richieste accettate precedentemente alla conversione in legge del decreto, verrà in ogni caso corrisposto il reddito di cittadinanza per almeno sei mesi,

Alla Camera dei deputati, il Gruppo Forza Italia ha presentato emendamenti migliorativi che sono stati però accolti solo eccezionalmente e in ridottissima parte: l'emendamento per cui si deve denunciare non solo il valore del patrimonio immobiliare posseduto in Italia ma anche quello posseduto all'estero, l'emendamento che specifica che il reddito di cittadinanza è compatibile anche con l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata ed infine quello che prevede il termine entro cui adottare il decreto ministeriale che disciplina il contributo INPS a copertura dei periodi contributivi scoperti per i lavoratori Altri emendamenti sono stati invece assorbiti, così come era successo in sede di prima lettura in Senato, per esempio l'aumento dei limiti del patrimonio immobiliare per i nuclei familiari con componenti disabili. Coerentemente con la nostra attenzione verso le fasce più deboli della popolazione abbiamo presentato fin dall'inizio degli emendamenti a favore delle persone con disabilità e dei nuclei familiari più numerosi,

La maggioranza ha voluto di fatto essere impermeabile alle molteplici proposte migliorative della minoranza e non ha dedicato attenzione e risorse a coloro che ne hanno veramente bisogno, a quanti hanno difficoltà anche ad accedere all'iscrizione perché in effettive condizioni di disagio sociale e che questo provvedimento rischia invece di escludere. Altro che abolire la povertà! Finalmente alla Camera dei deputati è stato posto rimedio, anche su nostra sollecitazione, ad una grave lacuna preesistente, escludendo l'erogazione del reddito di cittadinanza a chi sia stato sottoposto a misura cautelare personale o abbia avuto condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta, sempre che qualcuno in questa situazione non abbia già provveduto a fare richiesta del beneficio e, per via della norma transitoria che ricordavo prima, possa quindi percepire il reddito per i famosi sei mesi, salvo poi magari restituirvelo. Il provvedimento, da un lato, mira a sostenere i poveri, dall'altro, pretende di avviare i disoccupati alla formazione e all'inserimento nel mondo nel lavoro. Chi dovrebbe principalmente prendere in carico queste attività sono i centri per l'impiego e i Comuni, anche se i Comuni non sono pronti per le attività loro assegnate da questo provvedimento. Si tratterà infatti per loro di un onere enorme, che intaserà letteralmente la loro attività amministrativa e che dovrà essere fronteggiato con risorse proprie - già troppo scarse, soprattutto per i Comuni medio-piccoli - nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Ma sapete quanti Comuni hanno a disposizione questi fondi e in che misura? Colleghi della Lega, preparatevi bene, ma molto bene, a spiegare tutto ciò ai vostri sindaci nel territorio

Per quanto riguarda poi i centri per l'impiego, avevamo detto fin dall'inizio che non potevano essere pronti ed efficienti per svolgere tale attività e adesso siete stati costretti a prenderne atto; troppo tardi. Avete cercato di metterci una toppa, riscrivendo tutto l'articolo 12 per inserire il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, demandandolo tra l'altro ad un ennesimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tutto ciò, però, doveva essere già predisposto e attuato prima dell'avvio, non solo dell'erogazione, ma anche della richiesta stessa, anzi ben prima. Invece non vi è stato un approccio lungimirante, ma abborracciato e, soprattutto, vincolato ai termini della campagna elettorale delle elezioni europee, perché questo è il tema vero. modo, non è stato effettuato un confronto con le Regioni e gli enti preposti nei tempi dovuti, ma solo dopo aver già predisposto il decreto-legge. Vi avevamo anche detto che non si possono prevedere le assunzioni in massa dei cosiddetti *navigator* da dedicare ai centri per l'impiego in modo approssimativo, senza una progettualità. Ecco allora che le assunzioni sono demandate per un numero dimezzato rispetto a quello inizialmente previsto al 2020, mentre per ulteriori 4.600 unità al 2021. Ritardo negli accordi tra Stato e Regioni, ma anche mancanza di organizzazione e strutturazione, oltre che un'evidente scarsità di risorse. In sede di audizione si è presentato colui che sarebbe dovuto diventare il nuovo presidente di ANPAL e ANPAL Servizi, il professor Parisi, che quindi avrebbe da subito dovuto gestire il processo di ristrutturazione dei centri per l'impiego.

quindi evidente che non si abbiano le idee chiare né su come incrementare efficienza ed efficacia dei centri per l'impiego né su chi debba gestirne la riorganizzazione, senza considerare che intanto i tempi si allungano, i percettori di reddito non verranno presi in carico dagli enti preposti, mentre l'erogazione del sussidio proseguirà come puro assistenzialismo e il tutto avverrà in *deficit*. Non ce lo possiamo dimenticare: tutto tutto in *deficit*.

fanno veramente ridere rispetto al numero dei percettori del reddito di cittadinanza che dovranno essere controllati. Concludo dicendo che su quota 100 non sono state apportate grandi modifiche. Rimane una finestra limitata per poche persone e anche nel tempo, perché dura solo tre anni. Non è il superamento della legge Fornero. Noi ci aspettavamo di più. Rimane una misura costosa e ricordo che con il blocco dell'indicizzazione si tolgono soldi a quei pensionati che percepisco 1.200 euro al mese di pensione per pagare siffatta misura. tutto ciò è molto lontano dai programmi di Forza Italia e del centrodestra che gli italiani hanno votato l'anno scorso; i costi e le ripercussioni sul futuro non li avete considerati. erano e sono preponderanti gli obiettivi a fini elettorali, ma ricordate che anche e soprattutto dopo il 26 maggio le conseguenze della realizzazione del reddito di cittadinanza e di quota 100 vi metteranno di fronte

nell'*iter* parlamentare, nonostante le numerose e purtroppo sempre respinte proposte del Partito Democratico, il reddito di cittadinanza non muta nel suo impianto di fondo, confondendo sostegno al lavoro e contrasto alla povertà. In nessun Paese del mondo le due misure sono così confuse, perché il sostegno al lavoro abbisogna, oltre che di un sistema di accompagnamento alle persone, della promozione di un clima imprenditoriale che favorisca gli investimenti e crei nuove opportunità di lavoro, soprattutto nelle aree più deboli del Mezzogiorno. La lotta alla povertà porta con sé l'individuazione reale dei veri poveri, dei senzatetto, di tutti coloro che vivono spesso in famiglie a forte rischio di disagio sociale. Pur con tutti i limiti - lo dico - i Governi della XVII legislatura di Renzi e Gentiloni avevano individuato, da una parte il reddito, d'inclusione e, dall'altra, la costituzione, per la prima volta in maniera strutturale, di un'agenzia nazionale per le politiche attive, con la conseguente impostazione di una nuova una nuova impalcatura di diritti come - per esempio - l'assegno di ricollocazione per chi perde il lavoro. Secondo il Partito Democratico andava proseguita e rafforzata la strada intrapresa. Potevate anche chiamarlo reddito di cittadinanza - non ci saremmo soffermati su una questione nominalistica - ma bastava avere una impostazione giusta giusta del reddito di cittadinanza. La confusione, al contrario, recata in questo decreto-legge tra misure di sostegno al lavoro e contrasto alla povertà crea un mostro giuridico e il rischio concreto di non aiutare davvero i poveri veri, le disoccupate e i disoccupati, le persone con disabilità e in molti casi le donne. Fa male, come cittadina, ancor più che come rappresentante dei cittadini, rendersi conto che l'Italia farà un salto nel buio: è probabile che aumenteremo il debito pubblico e i nostri figli si troveranno domani a non poter prendere decisioni economiche perché stretti dalla morsa del debito, com'è già accaduto purtroppo nella nostra storia. libricino di Edmondo Berselli, purtroppo scomparso, che si chiama «L'economia giusta». A fronte dell'aumento del debito il reddito di cittadinanza lascerà indietro molte persone e famiglie davvero bisognose. E quota 100 rappresenta un intervento pensionistico a termine (fino al 2021) che, con la necessità dei due requisiti insieme (sessantadue anni di età e trentotto di contributi), non intercetterà lavoratrici e lavoratori più deboli e con carriere discontinue. Focalizzerò ora alcune modifiche apportate dalla Camera in tema soprattutto di intesa Stato-Regioni, disabilità, assunzioni, controlli, livelli essenziali delle prestazioni. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state introdotte molte novità, soprattutto in tema di intesa Stato-Regioni. Quanto tempo maggioranza ci avete fatto perdere in Commissione per chiedere una cosa che andava già inserita nel decreto-legge, ossia l'intesa Stato-Regioni, poiché sappiamo che sono materie di competenza regionale, alcune concorrenti. Avremmo dovuto dividerci sulle soluzioni politiche e non su una questione che andrebbe inserita. Vi faccio una domanda: perché non l'avete fatto prima? è presentato con un testo che già recepiva l'intesa Stato-Regioni? Sono molte le risposte: incompetenza - io difficilmente dico questo - o la mancata visione di uno Stato rispettoso dei vari livelli istituzionali,

Riteniamo che anche l'accordo politico con i livelli regionali, recepito nel testo approvato dalla Camera, sia stato molto importante. Ma in questo modo il comma 3 dell'articolo 12, da una decina di righe del testo iniziale, è diventato di due pagine nel testo modificato dalla Camera, aggiungendo i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*. Questo provvedimento, come molti altri del Governo, risente anche di una scrittura dei testi ridondante, noncurante dell'accessibilità delle norme, soprattutto quando esse si rivolgono a cittadine e cittadini maggiormente fragili.

che va avanti per somma di provvedimenti, purtroppo senza una visione d'insieme del Paese. Passiamo alla questione dei cosiddetti *navigator*.

Camera è stata apportata una modifica grazie all'intesa Stato-Regioni, e sono diventate 3.000 le persone con professionalità che andranno a fornire assistenza tecnica - questo dice l'intesa Stato-Regioni e il testo legislativo che oggi dovremo votare ma rimane il peccato originale: si immettono nei servizi per il lavoro in Italia 3.000 precari laureati, le cui modalità di selezione non sono ancora rese pubbliche, i quali dovranno essere formati sul campo presumibilmente da altri precari, che sono già operanti nell'ambito di ANPAL Servizi.

Nel corso del dibattito parlamentare il Governo ha risposto in maniera surreale e a tratti cinica - fatemelo dire, trattandosi di persone - alle nostre richieste di stabilizzazione di professionalità, che sono molto rare nel sistema italiano, adducendo motivazioni riferite al fatto che la situazione dei precari di ANPAL Servizi è responsabilità dei Governi della passata legislatura. È vero che sono ventidue anni che si accumula personale precario, avendolo ANPAL Servizi ereditato da Italia Lavoro,

dell'esame degli emendamenti, ma non c'è nulla nella scala di equivalenza che dia di più alle persone con disabilità. Si usa infatti una scala di equivalenza unica al mondo: non c'è da nessuna parte una scala di equivalenza che non dia di più a chi merita di più

dall'opposizione, senza fare sconti, perché ognuno dei nostri concittadini può avere il diritto di esigere quello che è previsto dalla legge e di esprimere i propri doveri.

ripercorso il dibattito tra le donne, nel femminismo, a proposito di salario e lavoro domestico. Ebbene, le donne scelsero il mercato del lavoro piuttosto che il salario del lavoro domestico. Analogamente al racconto di questa esperienza dobbiamo prendere ad esempio la vita delle donne e il loro desiderio di costruire una società di persone libere e solidali, con una politica che fornisca strumenti e opportunità per esserlo. che un reddito di cittadinanza senza percorsi di inclusione, i controlli al posto della responsabilità, le punizioni in luogo dell'accompagnamento e del sostegno, il reddito senza il lavoro e l'esclusione dei cittadini immigrati dagli aiuti sociali non siano le strade da percorrere per la nostra comunità anche questo il discrimine politico tra destra e sinistra. Continueremo a stare sempre dalla stessa parte, quella che persegue la libertà dal bisogno e l'emancipazione delle cittadine e dei cittadini, sostenendo chi si trova in difficoltà in un contesto ampio di sviluppo di opportunità di lavoro

Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, onorevoli membri del Governo, oggi siamo impegnati a discutere uno dei tanti provvedimenti *spot* che questo Governo ha voluto proporci o, meglio, imporci. Capisco che la linea politica di una maggioranza si sostanzia in alcuni capisaldi, ma è anche vero che misure come il reddito di cittadinanza e le pensioni non possono e non devono essere imposte attraverso l'uso e l'abuso della decretazione di urgenza. Si tratta di misure che avrebbero necessitato di un'ampia condivisione parlamentare e, invece - come già avete fatto con la legge di bilancio - per superare divisioni interne alla maggioranza costringete il Parlamento, come al solito, prendere o lasciare, senza creare quella giusta interlocuzione con le minoranze parlamentari che serve a migliorare i provvedimenti normativi, a contemperare le esigenze della collettività, che magari voi non vedete o non riuscite a considerare. Avete dovuto modificare più volte i presupposti di accesso al reddito di cittadinanza e alla pensione perché - ormai gli italiani lo hanno capito - la coperta è corta e siete consapevoli che, in assenza di un sistema efficace di controlli, gli abusi e le truffe saranno all'ordine del giorno. State dando un reddito di furbizia, senza peraltro aiutare le vere sacche di povertà e indigenza. State togliendo valore al lavoro per dare valore a un falso reddito di cittadinanza, che non è quel reddito di cittadinanza che avete promesso in campagna elettorale. Continuate a non occuparvi dei veri problemi, ma lo fate benissimo soltanto in campagna elettorale o all'opposizione, cercando di essere credibili e poi al Governo non riuscite a fare un provvedimento che sia coerente con quanto dite in campagna elettorale. Non vi state occupando del lavoro che manca sempre di più in tutto il Paese e soprattutto al Sud e tra i più giovani. Non vi state occupando delle opere pubbliche bloccate, della carenza infrastrutturale, che è la causa della mancanza di occupazione, soprattutto nel Centro-Sud. Non vi state occupando di quelle opere strategiche che costituirebbero un volano di sviluppo economico: l'alta velocità

Non volete che la ricchezza arrivi in Italia e al Sud e dal Sud; preferite l'assistenzialismo. Non volete completare la statale 106, che riguarda quattro Regioni, che non è percorribile. Non volete supportare gli aeroporti, che sono la prima fonte di ricchezza turistica di ogni Paese. Avete abbandonato le aziende agroalimentari al loro triste destino e saranno schiacciate dalla concorrenza e dalla contraffazione internazionale.

oppure di un vero sostegno alle famiglie che non hanno lavoro, di un vero reddito dignitoso e non di questo falso reddito. e non di questo falso reddito. Proprio sul reddito di cittadinanza Grillo è andato in Calabria a fare il suo spettacolo e ha offeso tutti i calabresi dicendo che sono 'ndranghetisti o lavorano in nero perché non hanno fatto la domanda per il reddito di cittadinanza in un paese che ha meno di mille anime. Non è giusto scherzare con qualcosa di così importante che offende la dignità di una Regione intera. Avete promesso miliardi per il reddito di cittadinanza per arrivare poi, forse, a 7 miliardi. Ecco perché non bastano le risorse. Colleghi della Lega, non potete accettare qualcosa di così inutile per i più bisognosi. Questo finto e demagogico decreto-legge, che non è un sussidio, non sarà mai un lavoro e addirittura rischia di trasformarsi in un meccanismo di distruzione del lavoro vero e di incentivazione al lavoro nero. Cari colleghi della maggioranza, ritornate con i piedi per terra. State guidando il Paese - e vorrei che lo dicesse anche De Falco - come Schettino ha guidato la Concordia: risalite sulla nave e salvate gli italiani.

Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentante del Governo, oggi licenziamo definitivamente, con ferma convinzione, la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, che reca disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e pensioni. Rispetto al testo già approvato in quest'Assemblea, la Camera dei deputati, in estrema sintesi, ha aggiunto ulteriori tutele per le famiglie al cui interno vi siano disabili e figli minori; aumentato i casi di sospensione o perdita definitiva del reddito di cittadinanza per alcune fattispecie di reati e condanne penali; ha soppresso il limite di quarantacinque anni per poter riscattare le annualità dei corsi di studio universitario. È previsto un incremento del personale preposto a verifiche e controlli sui richiedenti il reddito di cittadinanza. Quest'ultima è una misura unica e innovativa di contrasto alla povertà, alle diseguaglianze e all'esclusione sociale con ricerca attiva del lavoro. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da una o più persone di età pari o superiore a sessantasette anni si chiama pensione di cittadinanza. Con diversi emendamenti si è voluto evitare la possibilità che ci fossero richiedenti tentati dal dichiarare il falso pur di ottenere il suddetto beneficio, magari nell'impossibilità, da parte dei preposti al controllo, di verificare la veridicità delle dichiarazioni, come invece è possibile fare nei confronti dei nostri concittadini italiani ed europei. Sembra che ci siano persone desiderose di fare profitti e che taluni avvocati, tifosi dell'invasione dell'Italia, stiano affilando le loro armi per estendere questo beneficio indistintamente a tutti gli stranieri presenti nel Poiché sono stati acclarati più di 5 milioni di italiani in povertà assoluta, e le risorse economiche e finanziarie sono limitate, auspico che si comprenda quali siano le effettive intenzioni del legislatore e l'impossibilità materiale di poter mantenere tutti i diseredati che ci hanno già invaso.

I lavoratori privati che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2018 potranno ritirarsi dal lavoro già dal primo aprile; chi li raggiungerà successivamente potrà andare via tre mesi più tardi e la finestra è trimestrale. I lavoratori pubblici avranno invece finestre di sei mesi, con un preavviso di altri sei, e potranno lasciare il lavoro dal primo agosto. Per evitare disservizi nel mondo scolastico, i lavoratori della scuola, invece, dovranno aspettare il 28 febbraio di ogni anno per poter andare in pensione all'inizio del successivo anno scolastico o accademico. Tutti coloro che optano per la cosiddetta quota 100 - e finora è stata richiesta già da 100.000 lavoratori non potranno cumulare l'assegno con redditi da lavoro superiori a 5.000 euro annui fino al raggiungimento dei sessantasette Inoltre, il loro assegno pensionistico sarà più leggero, stante il versamento di minori contributi. Per favorire e stimolare il ricambio generazionale tra lavoratori anziani e giovani, la legge di conversione prevede lo sviluppo di una formula già esistente ma poco utilizzata finora. Le imprese in crisi o con esuberi potranno utilizzare i fondi di solidarietà di settore per consentire l'uscita con tre anni di anticipo rispetto a quota 100 (a cinquantanove anni e con Il fondo, con oneri a carico delle imprese, pagherà l'anticipo pensionistico fino al raggiungimento dei requisiti per quota 100. La novità è che le imprese non devono pagare anche i contributi per gli anni mancanti alla pensione. Il provvedimento oggi in esame si è reso necessario alla luce degli effetti distorsivi e devastanti della cosiddetta legge Fornero nei confronti del mercato del lavoro e dell'aumento sempre più preoccupante della disoccupazione giovanile. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo allungamento dell'età pensionabile per adeguarla alla speranza di vita dei lavoratori. La legge Fornero col tempo è diventata una diga di contenimento a un grosso bacino di lavoratori da tempo in età pensionabile, che la percepiscono sempre con maggiore insofferenza, in particolar modo nella pubblica amministrazione, dove il blocco del *turnover*, abbinato al prolungamento dell'età pensionabile, ha aumentato l'età media dei lavoratori a esageratamente elevata rispetto alla media europea. Al fine di ovviare a questo problema si è già intervenuti con il cosiddetto provvedimento concretezza che, sbloccando il *turnover* e consentendo un rapporto paritario fra lavoratori in entrata ed uscita, permetterà sicuramente un significativo e auspicato ricambio generazionale attraverso l'assunzione di giovani che sostituiranno i lavoratori che andranno in pensione. Quota 100 continua convintamente in questa direzione e nei prossimi tre anni cercherà di far defluire dal collo di bottiglia un po' di lavoratori, così da rendere successivamente più agevole il raggiungimento del vero obiettivo che si è posto questo Governo: quarantuno anni di servizio indipendentemente dall'età. Nel lavoro privato probabilmente non ci sarà di sicuro un ricambio paritario, ma si è voluto contribuire al ricambio generazionale fornendo alle aziende un impulso positivo che può renderle economicamente più forti, competitive e appetibili sul mercato del lavoro. Poiché questa opportunità è stata già accolta favorevolmente da 100.000 lavoratori in possesso di tali requisiti, possiamo affermare che avrà un impatto positivo sul mondo del lavoro; infatti, ci troviamo nella condizione di ribadire con forza che si può stimolare e sostenere il passaggio generazionale. Data l'età di molti lavoratori ancora in servizio si può dire che i nonni stanno lasciando il posto di lavoro ai figli;

un forte impulso anche per le natalità. Quota 100 è una facoltà volontaria, un modo aggiuntivo per accedere alla pensione insieme a tutti gli altri accessi ordinari già previsti o regolati dalla disastrosa riforma Monti-Fornero. Pertanto, si potrà continuare ad andare in pensione utilizzando indifferentemente sia la Fornero, sia quota 100, l'APE social, la pensione di anzianità, l'opzione donna o i provvedimenti previsti per i lavoratori precoci e quelli per le attività particolarmente usuranti. Fra le norme che stiamo approvando si prevede che l'INPS effettui un monitoraggio mensile per l'anno 2019 e trimestrale negli anni seguenti

disciplinano inoltre la riforma della *governance* dell'INPS, l'ente che gestisce le pensioni e l'assistenza, e quella dell'Inail, l'Istituto per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro. Dispone il passaggio da una gestione accentrata nelle mani del presidente a una collegiale «senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». In questi enti verranno ripristinati i consigli di amministrazione che erano stati aboliti molti anni fa, che saranno composti da cinque membri di nomina governativa, compreso il presidente. Oggi è un giorno speciale perché finalmente le Lega mantiene la promessa di scardinare la legge Fornero fatta in campagna elettorale. *(Applausi dal

colpendo i lavoratori italiana in maniera vigliacca, subdola e ingiusta, giustificando gli interventi come necessari e urgenti e facendo cassa a spese dei pensionati e di chi stava andando in pensione. Sono storie di questo Paese anche i miliardi di aumento del *deficit* pubblico che il Governo Monti ha prodotto e aggiunto sulle spalle dell'Italia. Quota 100 è un esercizio di coerenza per la Lega, che sancisce ufficialmente la fine di una stagione di supina obbedienza alle leggi calate dall'alto e dettate dall'alta finanza europea

Abbiamo così cercato di mitigare gli effetti punitivi di quella legge che, dall'oggi al domani, ha innalzato repentinamente l'età anagrafica di accesso alla pensione e allungato di parecchi anni la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed eliminato quella di anzianità.

Secondo la mia opinione, l'INPS dovrebbe essere scorporata tra assistenza e previdenza come negli altri Paesi europei: si farebbe finalmente luce sull'entità dei contributi versati dai lavoratori, che dovrebbero essere utilizzati esclusivamente

rappresentanti del Governo e colleghi, è un provvedimento, questo, che ha creato grande inquietudine anche all'interno del nostro movimento, perché abbiamo la consapevolezza

Tutto questo arriva alla vigilia di un appuntamento elettorale molto importante, quello delle elezioni europee del mese di maggio, per il quale credo ci sia un particolare interesse da parte delle forze politiche.

È un problema reale, quello della povertà in Italia. Sono milioni gli italiani in queste condizioni. La Lega aveva fatto una promessa iniziale. Quando

in oggetto, ci rendiamo immediatamente conto che 241.000 nuclei familiari che beneficeranno del reddito di cittadinanza sono composti da persone che provengono da Paesi stranieri. Dove è allora l'italianità? Lo dico agli amici della Lega:

di fronte a un provvedimento che darà aiuti, mance e sussidi a 241.000 nuclei familiari di stranieri. E ciò significa che 241.000 nuclei familiari di italiani non ne beneficeranno. Questo è un dato che dovrebbe assolutamente far

che non riuscirà a risolvere i problemi della povertà in Italia, perché la povertà - ricordiamo che sono princìpi elementari di economia - si aiuta attraverso la ricchezza. Non ho mai visto

quelle forme di impostazione economica di stampo marxista, che ancora albergano anche in questa Camera alta, ma soprattutto in Italia,

siete davvero convinti che tutta la platea a cui avete raccontato che andrà il reddito di cittadinanza effettivamente potrà beneficiarne. Credo che saranno molti di più gli scontenti e coloro che lo otterranno magari facendo i furbetti e, soprattutto,

Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, stiamo sicuramente parlando del provvedimento più importante per il Governo e la maggioranza che lo sostiene. La senatrice Catalfo lo ha addirittura definito di portata storica. Io per il momento non scomoderei la storia. Noi lo possiamo definire immediatamente rilevante anzitutto per l'impatto che genera sui saldi della finanza pubblica: oltre 40 miliardi di euro nel triennio, tutti finanziati ricorrendo al debito. Come rilevato dall'Ufficio parlamentare di bilancio - e questa è la prima misura strutturale che lo determina

rende strutturale l'incremento del debito scaricando sulle giovani generazioni, sull'Italia che produce, che lavora, che fatica gli oneri di questo incremento strutturale del debito.

Sì, lo diciamo con forza: abbiamo un'altra idea per contrastare le povertà, abbiamo un'altra idea per sostenere le politiche attive per il lavoro e abbiamo un'altra idea e un'altra visione anche di come sarebbe stato necessario intervenire sulle pensioni. Ripeto che di fronte a tutte le nostre proposte sono mancate le risposte da parte della maggioranza e del Governo; qualcosa a mio avviso di insostenibile, un'occasione sprecata, un errore politico della maggioranza, proprio perché attraverso il confronto cresce la qualità del dibattito e proprio perché solo attraverso il confronto si può allargare l'orizzonte e guardare un po' più avanti rispetto al triennio e un po' più in profondità nelle esigenze del futuro di questo Paese. Anzi, pur di fronte ad una terza lettura in Commissione bilancio, pur di fronte, quindi, ai limiti che la terza lettura determina nelle proposte emendative, noi ci siamo trovati a rivivere l'incubo della legge di stabilità, cioè ci è stata presentata una relazione tecnica e si pretendeva che, senza leggere quel documento, in pochi minuti, si arrivasse ad esprimere un parere. Peraltro, rinunciando a qualsiasi tipo di approfondimento, si determinano anche numerose ambiguità, che segnano una cattiva gestione politica del provvedimento, sia in prima che in seconda lettura alla Camera, sia in questa terza lettura al Senato.

e ci troviamo di fronte a relazioni tecniche che, nell'incertezza della platea, non rilevano oneri per la finanza pubblica. Se ci fosse stato un confronto di merito, avremmo potuto migliorare insieme il provvedimento, perché il Partito Democratico ha sempre sottolineato l'esigenza di incrementare le risorse per sostenere le povertà e per contrastarle nella dimensione territoriale. Se alzassimo un attimo lo sguardo e restituissimo una corretta centralità alla persona, ci accorgeremmo immediatamente che le politiche attive per il lavoro non sono sovrapponibili e non si possono confondere con le azioni necessarie per contrastare la povertà nella dimensione territoriale. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questo mi porta a dire con grande autorevolezza - lo ha ricordato molto bene prima la relatrice Parente

o 7.000 assistenti sociali da collocare nella dimensione territoriale per contrastare la povertà *(Applausi dal Gruppo PD)*rafforza in noi la convinzione che questo reddito di cittadinanza, così come è stato pensato, lascerà nella dimensione territoriale nuove povertà, povertà, ancora più forti, che rimarranno in solitudine nella dimensione territoriale perché non si è voluto rafforzare la presa in carico della povertà, che può venire solo nella dimensione territoriale. Dovevamo assumere un assistente sociale per distretto, dovevamo formarli in relazione alle nuove dimensioni sociali del fenomeno, che è molto complesso e molto diverso, lo abbiamo ricordato più volte. Non necessariamente chi è povero può trovare un lavoro e non necessariamente un disoccupato è povero: sono due casi diversi, due persone differenti, che probabilmente hanno bisogno di due azioni completamente distinte. Ecco perché era giusto incrementare le risorse per sostenere la povertà, così com'era giusto, d'altra parte, ridare centralità alle politiche attive attraverso la riforma del sistema dei centri per l'impiego. Queste azioni sono state confuse e l'esito (a proposito del non richiamare la storia) a mio avviso sarà negativo. Il tempo sarà galantuomo e dimostrerà gli effetti di questa misura. Signor Presidente, non è con l'ideologia del passato

non dire che si abolisce la Fornero, perché non è vero. Rispetto allo scalone che dovremmo recuperare tra tre anni, infatti, probabilmente chi sarà al Governo non disporrà delle risorse sufficienti per eliminarlo di fronte al contesto macroeconomico che si sta consolidando. Ecco perché diciamo con forza che questo è un provvedimento ideologico; utile a un'ideologia, ma probabilmente sbagliato nel merito al fine di garantire un futuro migliore alla crescita economica del nostro Paese. ripeto - che il tempo sarà galantuomo e ci auguriamo che si torni a pensare al futuro e alle giovani generazioni e non alle elezioni. Grazie.

ma nello stesso tempo mantenendo la nostra caratteristica: quando si votano o discutono le leggi, pensiamo sempre di fare qualcosa nell'interesse dell'intera popolazione del nostro Paese

è maggiormente avvertita dalle famiglie in cui vi sia un disabile. Vi ha ricordato la collega Toffanin che avete

volontariamente all'esecuzione della pena». Vi rendete conto dell'assurdità? In un provvedimento che si regge esclusivamente sul rapporto di fiducia

sua tecnica. Una parte della maggioranza non riesce immediatamente a percepire quali sono le correzioni che non hanno intento di contrapposizione politica. Quando presentai la suddetta correzione, che aveva una sua giustificazione dal punto di vista costituzionale,

onorevoli colleghi, finalmente oggi l'*iter* parlamentare di questo provvedimento cardine della manovra di bilancio per il 2019 arriva al suo ultimo voto. Finalmente oggi discutiamo del testo definitivo, così come ritoccato, rivisto e migliorato dal Parlamento. Sono orgogliosa di essere stata partecipe della buona riuscita di questo provvedimento che restituisce finalmente agli italiani quei diritti che erano stati negati in particolare a partire da quel fatidico 2011. Un provvedimento che da un lato restituisce la possibilità di anticipare la pensione a decine di migliaia di lavoratori e, dall'altro, aiuta quei cittadini in difficoltà economica, magari disoccupati, magari occupati ma con entrate insufficienti, a trovare un posto di lavoro con dignità. lavoro con dignità. Personalmente, il discorso sul reddito di cittadinanza non mi ha mai appassionata e invece il grande lavoro parlamentare ha fatto sì che si arrivasse ad una formulazione che riesce a legare strettamente il contributo contro la povertà all'inserimento e al reinserimento lavorativo, evitando al meglio l'accesso al beneficio per i cosiddetti furbetti. Penso ai requisiti di residenza, ai controlli sui beni immobiliari, al monitoraggio previsto sui cambi di residenza avvenuti a partire dal 1° settembre 2019 e, per evitare discriminazioni tra italiani e stranieri, arriva la cosiddetta norma Lodi con la quale anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sono tenuti a produrre l'apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana. Sono esclusi dal reddito di cittadinanza coloro che sono sottoposti a misura cautelare personale o coloro che sono stati condannati per talune fattispecie delittuose. Insomma, tutto converge in un provvedimento il cui fulcro è il lavoro. Con quota 100 non so se si creeranno più posti di lavoro di quanti beneficeranno dell'anticipo pensionistico, ma un dato è certo: si creeranno nuovi posti di lavoro. Su quota 100 già tante parole sono state dette. Voglio ricordare che si tratta di una lotta ormai storica della Lega. Tutti i colleghi del mio Gruppo ricorderanno le giornate trascorse sotto i gazebo a raccogliere le firme per l'abolizione della legge Fornero. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Io in prima persona, nella mia Piossasco, ne ho raccolte tante di firme. Noi sì che abbiamo toccato con mano il disagio di una vasta fascia di lavoratori ingiustamente penalizzati ed oggi, con quota 100, abbiamo trovato la formula migliore per superare la legge Fornero, la formula per raggiungere l'obiettivo l'obiettivo di dare la possibilità ai lavoratori, che tanto hanno già contribuito al tessuto produttivo del nostro Paese, di andare in pensione fino a cinque anni prima.

fa un lavoro appagante, non usurante, ma stressante, perché sempre in viaggio. Ha qualche problema di salute e, con la legge Fornero, avrebbe dovuto obbligatoriamente attendere marzo 2021 per andare in pensione. Ebbene, signori, Walter il prossimo mese di maggio andrà in pensione: dice che imparerà a volersi bene e finalmente potrà dedicarsi di più alla sua famiglia. Grazie.

credo che la parola d'ordine che è rimbalzata in tutti gli interventi fatti dall'opposizione, sia da parte nostra che da parte del Partito Democratico, fa leva sul concetto di confusione. cui stiamo discutendo è soprattutto confusivo e voglio spiegarmi, perché è proprio dalla chiarezza che si sarebbe potuta fare e che invece non si è voluta fare che dipenderanno poi l'effettiva applicazione e i risultati che si potranno o meno raggiungere grazie a questo provvedimento. La prima confusione si fa mettendo insieme le politiche per la povertà, che vanno incontro a situazioni e a contesti in cui i bisogni delle persone sono, per esempio, quelli legati alla salute (penso alla grande categoria delle disabilità, dei malati cronici e con malattia rara), e con malattia rara), con quelle rivolte a coloro che non hanno condizioni concrete di formazione e di competenze raggiunte, con un profilo formativo, non solo scolastico, ma anche professionale e di apprendistato. Per queste persone le misure avrebbero dovuto avere un sapore totalmente diverso: avrebbero dovuto chiamare in causa in modo molto più sostanziale quello che è

quali competenze maturano effettivamente i nostri giovani dopo la scuola media superiore, dopo un percorso di laurea, dopo un *master* e un dottorato. Perché non trovano lavoro? Perché persone con altissimi profili di competenza non trova lavoro? C'è la possibilità che forse queste competenze non siano concordate o in qualche modo armonizzate adeguatamente con le attuali richieste del mondo

il passaggio alla Camera ha avuto un valore incrementale sotto il profilo della cultura del sospetto: ho sentito parlare di furbetti. È possibile,

mette i ragazzi in condizione di essere non soltanto formati, ma anche formati in funzione del lavoro. È chiaro che i famosi 780 euro sembrano tantissimi se li confrontiamo con i 500 euro che molte persone che lavorano nei *call center* possono percepire

Mi permetta anche di fare riferimento, per quanto riguarda quota 100, a una domanda che sembra occupare l'orizzonte delle speranze, da un lato, e della diffidenza, dall'altro: davvero per ogni persona che uscirà ci sarà una nuova persona che vi entrerà? Mi chiedo inoltre se siamo sicuri che alla saggezza e all'esperienza accumulata nel tempo potranno rispondere le nuove competenze, sia pure quelle maturate nel campo della digitalizzazione, capaci di garantire anche a tutta la grande politica del pubblico impiego un rinnovamento del lavoro burocratico, che oggi come oggi è veramente un cimitero degli elefanti? Siamo sicuri che da questo possa derivare un effettivo incremento nella qualità dello sviluppo del Paese o avremo semplicemente appesantito la nostra macchina burocratico-amministrativa, togliendo speranza e perdendo una grande opportunità? Concludo dicendo che resta per me un elemento di grande dispiacere pensare che i più poveri dei poveri, quei poveri senza dimora e senza residenza, non potranno nemmeno aspirare

sperimentale povertà e miseria di queste persone. Non aver pensato a loro è un ulteriore *vulnus* del decreto-legge in

oggi noi del Movimento 5 Stelle siamo emozionati e felici perché stiamo per approvare definitivamente un complesso di norme che contribuiranno concretamente a far vivere meglio tanti milioni di italiani che la cattiva politica aveva dimenticato o ignorato e che noi, invece, abbiamo messo al centro della nostra azione. Stiamo finalmente per approvare un provvedimento che è una delle colonne portanti della proposta politica del MoVimento 5 Stelle; un provvedimento che ha lo scopo di contrastare l'impoverimento progressivo di milioni di italiani che non trovano lavoro o che, pur lavorando, si trovano sotto la soglia di povertà essendo sfruttati e vessati; un provvedimento che ha lo scopo di migliorare le politiche attive per il lavoro, di aumentare le pensioni e di superare la sciagurata legge Fornero. Ci arriviamo oggi dopo esserci contrapposti per anni alle altre forze politiche su tali tematiche, perché il MoVimento 5 Stelle ha proposto il reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero sin dal suo ingresso in Parlamento nel 2013. Questa contrapposizione politica è stata totale, ed è stata ribadita ieri ed oggi dai colleghi delle opposizioni. come loro, descrive alcuni milioni di italiani come fannulloni, come truffatori, come gente che rimarrà sul divano e percepirà comodamente il reddito di cittadinanza. E c'è chi, come noi del MoVimento 5 Stelle, vuole aiutare questi nostri connazionali colpiti dalla crisi economica, dalle politiche di austerità e dalle disuguaglianze che dal 2011 ad oggi sono aumentate a dismisura. Soprattutto, c'è chi, come noi del MoVimento 5 Stelle, vuole dare attuazione, dopo settant'anni, all'articolo 38 della nostra amata Costituzione, il quale statuisce che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». Ripeto: mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria. La risposta a questo problema è nel reddito di cittadinanza e nelle politiche attive del lavoro, che noi oggi approviamo definitivamente. In questi ultimi anni e mesi, e ancora oggi, si è palesata chiaramente la contrapposizione tra il MoVimento 5 Stelle, che vuole dare attuazione ai princìpi costituzionali, e alcune forze politiche e alcuni potentati economico-finanziari, che vogliono lasciare le cose come stanno, forse perché fa comodo tenere in condizioni di bisogno e di disperazione milioni di italiani a cui, magari, chiedere il voto e il sostegno a ogni tornata elettorale. *(Applausi Tra l'altro, questa contrapposizione tra visioni politiche e socioeconomiche diverse si palesa per la verità ad intermittenza, perché in campagna elettorale invece eravate tutti a favore del reddito di cittadinanza. Sono indimenticabili, a questo proposito, le dichiarazioni di Berlusconi,

Per fortuna degli italiani, il MoVimento 5 Stelle è diverso, non dimentica gli impegni elettorali, anzi li mantiene, e in questo caso li tramuta in provvedimenti di legge in solo otto mesi di Governo. Il reddito di cittadinanza cambierà radicalmente la vita e il futuro di milioni di italiani che oggi soffrono, perché non sarà un sussidio assistenziale - come ancora oggi abbiamo sentito - ma sarà implementato da un sistema efficiente e articolato di politiche attive politiche attive per il lavoro, basato sui centri per l'impiego che saranno finalmente messi in condizioni di ben operare anche grazie alle migliaia di nuove assunzioni di operatori, a cui si affiancheranno i *navigator* i *navigator* che prenderanno in carico i beneficiari del reddito di cittadinanza e li accompagneranno, passo dopo passo, fino al nuovo impiego. Inoltre, si realizzerà il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che sarà collegato al sistema informativo unitario dei servizi sociali, il che permetterà di interconnettere tutte le banche dati dati esistenti, in modo che di ogni lavoratore si conoscano la formazione e le competenze, da mettere a disposizione delle aziende presenti sul territorio nazionale. L'investimento complessivo nelle politiche attive del lavoro sarà di circa 2 miliardi nel biennio 2019-2020. Questi interventi aiuteranno a colmare il *gap* che in questo settore esiste tra il nostro e gli altri Paesi europei, che è figlio di politiche del lavoro sbagliate dei precedenti Governi. A titolo di paragone, si pensi che nei centri per l'impiego di Germania e Francia lavorano rispettivamente 100.000 e 54.000 addetti: sono numeri enormi rispetto ai nostri attuali (8.000).

A volte capita, infatti, che l'offerta di lavoro esista, ma che non venga soddisfatta perché non sono stati mai approntati strumenti per incrociare domanda e offerta. Basti pensare che, attualmente, i centri per l'impiego non comunicano tra loro e che, addirittura, alcuni sono sprovvisti di un proprio sito Internet. Ma tutto questo cambierà. La riforma strutturale che oggi approviamo definitivamente aiuterà a rimettere nel circuito della formazione e della ricerca attiva del lavoro anche una parte di quegli oltre 3 milioni di inattivi che, da anni, non cercano più fattivamente E questo aspetto importantissimo della nostra riforma, ossia il previsto afflusso di questi scoraggiati e inattivi presso i centri per l'impiego, permetterà di rivedere al rialzo il tasso di partecipazione alla forza lavoro che, per il metodo di calcolo adottato in Europa, contribuirà alla crescita del PIL potenziale, il che migliorerà i conti pubblici. Del resto, oltre a queste considerazioni, ce ne sono tante altre di natura strettamente economica, che dovrebbero far riflettere chi, continuamente, parla di mercato, di liberismo e di crescita. Infatti, continuare ad avere 5 milioni di poveri, che inevitabilmente rimangono ai margini della società, costituisce un vero e proprio danno economico per l'intero Paese, perché questi nostri connazionali sfortunati non hanno potuto contribuire, fino ad oggi, al progresso e al benessere collettivo e, ad esempio, si sono ammalati in misura maggiore rispetto agli altri e quindi hanno usufruito in misura maggiore del Servizio sanitario nazionale, costituendo dunque un ulteriore costo per lo Stato. In definitiva, i vantaggi che porterà al nostro Paese il reddito di cittadinanza non li vede solo chi si copre gli occhi, perché non li vuole vedere. Per ciò che riguarda la famigerata legge Fornero, in campagna elettorale noi del MoVimento 5 Stelle avevamo preso l'impegno di superarla, istituendo la favorendo il ricambio generazionale, liberando posti di lavoro per i giovani e, in tal modo, ringiovanendo e migliorando le competenze della forza lavoro. In buona sostanza, con il provvedimento in esame si compie il primo passo per risolvere quello spaventoso conflitto generazionale, che ha costretto migliaia di ultrasessantacinquenni a continuare a lavorare e che ha causato la disoccupazione o l'emigrazione di centinaia di migliaia di giovani. Grazie al provvedimento in esame, fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle, un milione di lavoratori nel prossimo triennio potrà anticipare la pensione fino a cinque anni rispetto ai requisiti della legge Fornero. Concludendo, oggi non approviamo solo un provvedimento di legge atteso da anni da milioni di italiani che soffrono. Oggi arriva a compimento una parte importante di un percorso politico, un pezzo delle nostre vite di attivisti e di portavoce del MoVimento 5 Stelle, che valeva la pena di essere vissuto. *(Applausi Grazie Signor Presidente, membri del Governo, inizio il mio intervento con una convinzione: il *welfare* è una delle conquiste più importanti e più nobili dell'azione politica dell'ultimo secolo. però da stare attenti, perché le attuali politiche internazionali, spesso ispirate a un processo di radicale liberalismo e di globalizzazione senza umanesimo,

di tante donne, laureate e non, di commercianti, che per loro sfortuna hanno dovuto chiudere la loro attività per colpa della crisi, di tanti professionisti ormai incapaci di continuare la propria attività, di tanti lavoratori di mezza età che hanno perso il loro posto di lavoro. Con queste categorie anche io mi confronto giornalmente e, ahimè, la frustrazione più grande è quella di non poter offrire loro una risposta immediata e una soluzione dei loro problemi. Per alleviare questo disagio occorre sì continuare ad individuare dei metodi per rafforzare il *welfare* ma, cari colleghi del Governo, serve soprattutto creare occupazione, lavoro, sviluppo e investimenti strategici. I provvedimenti occasionali come il reddito di cittadinanza limitati nel tempo e assolutamente disancorati da ogni prospettiva di crescita purtroppo non offrono alcun rimedio. Nel merito della proposta del reddito di cittadinanza va detto innanzitutto che potrebbe essere destinato a una platea assolutamente inferiore rispetto a quanti ne avrebbero bisogno. In effetti, la discordanza tra i dati dell'INPS e quelli del Governo sono sotto gli occhi di tutti, ma voi, colleghi del Governo, non ne avete assolutamente preso atto. Siamo di fronte a un vero bailamme, con il rischio che ampie fasce della popolazione in stato di povertà non siano raggiunte da questa misura.

che a un disoccupato beneficiario del reddito di cittadinanza - penso sempre alla mia Regione Calabria - vengano offerte in diciotto mesi non una o due, ma ben tre proposte di lavoro congrue?

vi siete impegnati ad assumere a tempo determinato dei commessi e dei lavoratori (che sono i *navigator*), ma non vi siete in alcuna maniera

il rischio è che cento rischi di diventare l'età di pensionamento della nuova generazione perché, purtroppo, queste scelte scellerate hanno un prezzo economico altissimo che pagheranno, in modo particolare, le future generazioni. *(Applausi

Come premessa vorrei dire che farò finta che siano rispettate le condizioni ideali, come succede in fisica e, cioè, che i percettori siano realmente poveri, non ci siano truffe, finti licenziamenti e altre gabole di questo tipo. *(Commenti Detto questo, un'erogazione di questo tipo dovrebbe essere in teoria un reddito di base e, come tale, totalmente svincolato da richieste di natura lavorativa. Questo è lo spirito e su un intervento di questo tipo sarei assolutamente d'accordo.

sui profitti, sul patrimonio o sui grandi redditi. A prescindere dal fatto che possa essere d'accordo o meno con questa filosofia di tassazione e di redistribuzione, questo principio non viene rispettato. rispettato. Lo paga, quindi, la platea indistinta dei contribuenti perché il maggior debito e gli oneri sul debito sono pagati dalla collettività indistinta. luogo, non è una misura che genera ricchezza purtroppo. Anche in questo caso la matematica, per fortuna, viene sempre ad aiutarci. La prima stima che è uscita dice che questa misura - che non si chiama neanche «reddito di cittadinanza», perché non andrà solo ai cittadini italiani, come era stato promesso per molto tempo - produrrà un incremento del PIL di circa lo 0,2 per cento, a fronte di un'erosione potenziale del PIL dello 0,4-0,5, perché il rapporto tra le risorse investite e il PIL è tra lo 0,4 e lo 0,5. Ciò significa che c'è un impoverimento netto nazionale che vale circa lo 0,2-0,3 per cento del PIL, e questo è un numero. Quindi, il famoso moltiplicatore keynesiano, che è stato invocato per dire che questa manovra avrebbe generato più di quanto costava,

perde. Purtroppo - e dico purtroppo, perché personalmente sono favorevole a un reddito incondizionato - questa misura comporta un impoverimento netto nazionale, perché gli acquisti, supponendo naturalmente che ogni percettore faccia un acquisto di tipo etico, verranno dirottati (essendo percettori a basso reddito) su beni di prima necessità: beni di consumo, non beni durevoli. I beni di consumo, come sappiamo, sono per la maggior parte di importazione. Quindi, ogni volta che compreremo qualcosa che è un bene di importazione ci sarà un deflusso netto di capitali verso l'estero. Se anche lo spirito era «compra italiano», purtroppo una persona che ha poco reddito disponibile va a comprarsi qualcosa che costa poco; quindi, deflusso netto di capitali. A tal proposito apro un inciso sul controllo di eticità degli acquisti. Supponendo che idealmente si fosse fatta una cosa di questo tipo, a me purtroppo fa molto pensare alla famosa tessera annonaria: il diritto ad acquisire un paniere di beni e servizi che sono stabiliti a livello etico nazionale. Colleghi, questa non è una bella cosa; non lo è per niente. Non mi soffermo sui controlli, perché ovviamente la mole dei controlli insufficienti che vengono messi in campo fa capire come la trasposizione al reale di un provvedimento ideale raramente può funzionare. Ho già fatto l'esempio: posso prendere questa tessera, metterla in una busta, spedirla a un parente che sta in Costa Rica; questa persona fa degli acquisti, la rimette nella busta, mi mette il contante, me la rispedisce ed è tutto regolare, perché non c'è neanche un controllo sulla localizzazione del pagamento. Si tratta di un altro aspetto importante di cui tenere conto. Faccio un brevissimo inciso - e concludo - su quota 100. Sono assolutamente d'accordo a qualunque provvedimento che consenta l'uscita anticipata dal mondo del lavoro; vorrei, però, che all'interno di questa Aula e nel futuro ci si ponesse il seguente problema: come vogliamo trasformare il sistema pensionistico italiano. Molto praticamente su cosa è basato il sistema pensionistico? Su una proiezione della durata residua mediana della vita. L'INPS fa questo tipo di calcolo e dice che se la vita mediana dura *tot* e si va in pensione a una determinata data, allora c'è uno sbilancio positivo per l'ente previdenziale, con la conseguenza che l'ente previdenziale si autosostiene. La quota 100, naturalmente, è una misura temporanea ma nel futuro, con l'aumento della vita media e mediana, la sostenibilità di un sistema pensionistico il problema di gente che dovrà lavorare

che il provvedimento oggi in esame, con particolare riferimento al reddito di cittadinanza, sia il più clamoroso caso di pubblicità ingannevole di questa legislatura - e forse anche di quelle precedenti - credo sia ormai chiaro a tutti. È chiaro anche agli italiani, visti i risultati elettorali che il MoVimento 5 Stelle sta conseguendo laddove, grazie alla pubblicità ingannevole del reddito di cittadinanza, soltanto un anno fa aveva conseguito percentuali bulgare. È pubblicità ingannevole, cari colleghi, perché basta una semplice calcolatrice per rendersi conto che 780 euro al mese con le somme stanziate dalla legge possono soddisfare soltanto 750.000 persone, mentre, ipotizzando una platea di 5 milioni di persone, come ha fatto il ministro Di Maio, il risultato sarebbe molto semplice: 133 euro a persona. Pubblicità ingannevole volta, come hanno già detto molti colleghi che mi hanno anticipato, a conseguire qualche voto in più alle prossime elezioni europee. se anche così non fosse, entrando nel merito, è evidente che si tratta di una misura che rappresenta un potente incentivo al lavoro nero. imprese (CGIA) di Mestre i lavoratori in nero oggi sono circa 2 milioni. È difficile immaginare che il reddito di cittadinanza non vada in gran parte anche a costoro. Ricordo che 4,2 milioni di contribuenti italiani percepiscono all'anno meno di 10.000 euro;

che rappresenterebbero l'offerta congrua secondo il provvedimento al nostro esame. Un soldato guadagna 850 euro al mese, un poliziotto guadagna dai 1.100 ai 1.200 euro al mese.

in vigore nel Paese. Esattamente il contrario di quello che state facendo voi. E che si tratta di una norma criminogena la riconoscete voi stessi. Come Come sancisce la Guardia di finanza, il 40 per cento delle dichiarazioni ISEE non sono veritiere. Ecco perché alla Camera hanno stabilito di assumere 100 funzionari della Guardia di finanza e 65 carabinieri per andare a controllare le dichiarazioni e le pratiche dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Avete messo nuovi agenti di polizia giudiziaria non a perseguire reati, non a contrastare la criminalità, ma a controllare le dichiarazioni ISEE e le pratiche dei beneficiari del reddito di cittadinanza perché vi rendete conto benissimo che state approvando una legge che determinerà migliaia di migliaia di persone a commettere dei reati. State facendo una legge per indurre la povera gente a commettere dei reati! Questo è ciò che state facendo, cari colleghi della maggioranza. Noi di Fratelli d'Italia avevamo detto che la strada era un'altra, quella di incentivare le imprese ad assumere e a creare lavoro vero, non assistenzialismo per lasciare la gente sul divano tutto il giorno. Avevamo proposto - e ce li avete respinti - 20.000 euro di decontribuzione per ogni nuovo assunto dalle imprese: così si sarebbe creato lavoro vero. Avevamo anche chiesto il raddoppio delle misere pensioni d'invalidità per coloro che hanno davvero bisogno, ma anche questo ce lo avete respinto. Avevamo chiesto il reddito di maternità per far sì che l'Italia non fosse l'ultimo Paese al mondo

è che sappiamo benissimo non solo che il reddito andrà a tantissimi furbetti, magari a discapito delle persone perbene, che ne avrebbero davvero bisogno, ma che vi è una cosa ancor più vergognosa: voi date il reddito di cittadinanza anche ai delinquenti,

di escludere dal beneficio tutti coloro che hanno conseguito condanne superiori ai due anni, è esattamente così. Anche la norma inserita dalla Camera, per cui sarebbero esclusi coloro che sono stati o sono sottoposti a una misura cautelare personale, è ridicola. ridicola. Non ci vuole un giurista per sapere che le misure cautelari oggi possono essere applicate soltanto in determinati e specifici casi (gravi indizi di colpevolezza, pericolo di fuga,

è la norma che state approvando ed è per questo che noi di Fratelli d'Italia non soltanto voteremo contro questo disegno di legge, ma da domani cominceremo a raccogliere le firme per il *referendum* abrogativo

cresce l'incertezza e aumentano quelle che prevedono un calo della produttività: è l'Istat che vi parla, dopo aver fotografato a colori

festeggiate la vostra organizzazione del consenso; aspettate con particolare attenzione le elezioni europee, convinti di poter festeggiare anche in quell'occasione.

Come e cosa rispondete alle imprese? Come e cosa rispondete ai giovani e ai disoccupati? Come e cosa rispondete al Sud del Paese, che piange lacrime di dolore? Con il reddito di cittadinanza, cioè con un sussidio: la peggior terapia

non è stata elaborata dal MoVimento 5 Stelle. Sarebbe troppo comodo, amici e colleghi della Lega. Questa è una terapia elaborata, costruita, costruita, pensata e studiata scientificamente dal Governo. Se le cose andranno bene, il merito sarà del Governo; se le cose andranno male,

C'era la possibilità di correggere un testo, secondo me inemendabile, ma ci siamo comunque sforzati e abbiamo esercitato un'attività emendativa costruttiva.

di una contraddizione in termini: non è possibile garantire dei livelli essenziali di prestazione e poi vincolarli alla compatibilità delle risorse.

è sempre più crescente la difficoltà di "sbarcare il lunario". E mortificate anche quelle famiglie all'interno delle quali ci sono bambini.

che ha elaborato una soluzione di questa portata. Non chiedetelo a me: chiedetelo alle associazioni, al terzo settore, se ho visto bene o ho visto male.

Quota 100 è una vera e propria lotteria, lotteria, che sarà pagata dalle future generazioni e - su questo potete stare tranquilli,

ho passato il tempo a raccogliere le firme e ad ascoltare le storie delle persone che sottoscrivevano la nostra proposta. Erano storie di persone normalissime, che avevano fatto dei programmi di vita e che vedevano gli stessi completamente distrutti. Quei programmi di vita

permettendo ai propri familiari di inserirsi nel mondo del lavoro, di continuare a lavorare, di rientrare dopo una maternità il prima possibile, insomma di fare una vita normale

noi cominciamo a cancellarne una grande parte e questo è un successo.

quali si legiferava soltanto con la decretazione d'urgenza (ovviamente sia a destra che a sinistra, ma questa era la modalità). Mi sembra che questa sia la prima legislatura durante la quale si usa molto meno la decretazione d'urgenza e questo penso sia un'altra risposta al collega Manca, il quale lamentava moltissimi aspetti: ricordo sommessamente che partiamo dai vostri risultati,

un sondaggio tra gli insegnanti, più che parlare bene della legge sulla buona scuola ci chiedono quota 100. Tutti quest'anno hanno continuato a chiederci quando avremmo portato avanti quota 100.

dopo le considerazioni di merito che il mio Gruppo ha ampiamente argomentato, consentitemi di aggiungerne alcune di carattere generale. Il disegno di legge al nostro esame avrà un impatto sia sulla vita degli italiani che sui conti pubblici. Lo avrà sulla vita degli italiani più poveri che noi per primi abbiamo sempre avuto a cuore (la carta acquisti l'ha inventata il Governo Berlusconi ed è bene ricordarlo sempre), ma l'avrà anche sulla vita di tutti gli altri italiani, perché le scelte di carattere economico o di politica economica non possono mai essere considerate neutrali. Non basta quindi dire che con il reddito di cittadinanza aiutiamo i poveri, come hanno affermato i due *Vice* *Premier*; la misura contenuta in questo disegno di legge ormai non può più essere venduta con gli argomenti della propaganda elettorale. Adesso ha numeri precisi

Si aiuteranno sicuramente un certo numero di famiglie, ma se ne lasceranno fuori molte altre, posto che le persone considerate povere in assoluto in Italia sono 5 milioni. Non si aiuteranno gli ultimi perché almeno un milione e mezzo dei veri poveri rimarranno esclusi da qualsiasi beneficio, come è stato ricordato in quest'Aula in un intervento precedente al mio dalla senatrice Binetti, che naturalmente - fuori da quest'Aula - da associazioni come la Caritas. A prendere il reddito ci saranno senz'altro i più scaltri, i più avveduti a districarsi in una misura che, come tutte quelle a forte vocazione assistenzialista, si presta ad essere aggirata. Si tratta di un intervento assistenziale dunque, che avrà effetti sociali simili a quelli creati sinora dalle false pensioni di invalidità, dal reddito garantito ai lavoratori socialmente utili e dall'accoglienza umanitaria accordata agli stranieri. Ma soprattutto va ricordato - e lo ripeto

parla di circa 241.000 stranieri, che potrebbero però essere 480.000 se venissero accolte le pronunce più volte ribadite ribadite da parte della Consulta per cui cinque anni sarebbe il limite del soggiorno di lunga durata, il che raddoppierebbe il numero degli stranieri. Dunque in questa legge vengono prima gli stranieri che si prenderanno più di un terzo degli assegni e lo stesso termine «cittadinanza», quindi, non sembra essere appropriato questa forma di sostegno al reddito. Soprattutto non può essere considerata una misura per l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro per mancanza di offerta di lavoro attraverso i centri per l'impiego e per la tortuosità burocratica del percorso richiesto. I centri per l'impiego - lo ribadisco oggi - sono assolutamente impreparati a gestire tutte queste pratiche e non hanno avuto il tempo necessario per riorganizzarsi. Il legislatore deve prima riorganizzare la macchina burocratica e solo leggi di questo tipo, non il contrario. Ma torniamo agli aspetti di finanza pubblica: nella legge di bilancio si sono creati due fondi ricorrendo a nuovo indebitamento per oltre 11 miliardi di euro per accogliere le misure previste per accogliere le misure previste con questo provvedimento. Mi avvio a concludere, Presidente, non senza ricordare che oggi, in quest'Aula, non avremmo dovuto parlare noi della Commissione lavoro ma avrebbero dovuto parlare i membri della Commissione bilancio e finanze. Infatti le stime che oggi riporta «Il Sole 24 Ore», che non sono sicuramente di questo giornale ma delle più autorevoli società

Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, molti economisti del passato come James Meade, Oskar Lange, anche conservatori come von Hayek, Milton Friedman e Karl Polanyi hanno sostenuto la necessità economica e sociale di uno strumento di sostegno al reddito nelle diverse varietà di sussidio sociale, di reddito garantito, di dividendo sociale, di reddito minimo. L'esigenza di uno strumento come il reddito di cittadinanza trova le sue basi nella Costituzione italiana agli articoli 3 quali si ritiene necessario l'intervento dello Stato nel rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Si stabilisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale dei poveri, degli indigenti e dei disoccupati. L'articolo 14 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce chiaramente il diritto al reddito minimo per garantire una vita dignitosa e ritiene utile combinare tale reddito minimo con incentivi all'integrazione nel mercato del lavoro. In periodi di crisi, come quella che ha colpito gran parte dell'Europa dal 2009 in poi, strumenti come il reddito minimo sono necessari per stabilizzare o almeno compensare il ciclo negativo, sostenere i consumi, la domanda aggregata e quindi l'economia, evitando anche e soprattutto l'esplosione della povertà. Questo però è ciò che è accaduto in quanto, in base ai dati Eurostat del 2016, l'Italia risulta essere il nono Paese per livelli di povertà

posto, ad indicare una bassa efficienza del nostro sistema sociale, appunto a causa dell'assenza di uno strumento di ultima istanza sociale quale il reddito di cittadinanza.

Questo indice di povertà ha continuato a crescere in maniera costante dal 2014, perché due lunghe recessioni hanno danneggiato il tessuto sociale del Paese. Il reddito di cittadinanza doveva essere istituito già da tempo, ma così non è stato. Il vecchio sistema probabilmente ha fallito: è questo che stiamo cercando di capire. In questo Paese non è mai stata data la giusta importanza al lavoro, ai lavoratori e alle famiglie, tutti temi di cui ci si è occupati solo marginalmente o durante le campagne elettorali. Il primo dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, collegato all'attuazione di tutti gli altri, è sconfiggere la povertà. Ciò significa che agire con strumenti di contrasto alla povertà, come il reddito di cittadinanza, è indispensabile per realizzare gli altri 16 obiettivi di sostenibilità, tra cui figurano una stabilità economica e la riduzione delle disuguaglianze. La bontà della nostra misura è confermata anche dall'indicatore BES, ossia dall'indicatore del benessere equo e sostenibile. Perdonatemi, io non parlerò del PIL perché il PIL non ci ha mai fatto sapere nulla della povertà che continua ad aumentare in Italia.

BES? Ci dice che il reddito di cittadinanza e quota 100, che è l'altro pilastro della nostra riforma, sono strumenti ad elevato potenziale di aumento del reddito *pro capite*, in grado di ridurre le disuguaglianze arginando la povertà assoluta. Sono state dette cose assurde: si manovra per i furbi, per gli scansafatiche. Io non riesco tranquillamente a vedere sul divano chi un momento prima sta cercando tra i rifiuti per trovare qualcosa da portare in tavola e queste cose le abbiamo viste tutti. Provate a dirlo poi a una famiglia che stenta ad arrivare a fine mese perché magari tutti e due i genitori sono disoccupati. Bisogna avere il coraggio, perché è molto facile parlare di furbetti dietro una telecamera o dietro uno schermo. Provate a dirlo in faccia a queste persone

i loro coetanei occupati si ferma al 3,5 per cento. Questo è un dato preoccupante, quindi uscite dal vostro guscio e guardate la realtà, confrontatevi con la gente, ascoltatela Noi siamo continuamente nelle piazze, tutti i sabati e tutte le domeniche, perché siamo cittadini tra i cittadini, perché li ascoltiamo, ascoltiamo il territorio. Parliamo quindi di benessere non di ben-avere o di profitto, perché noi facciamo riferimento a persone, individui che necessitano di cura; parliamo di cittadini che hanno dei diritti, come il diritto ad un lavoro e ad avere politiche attive efficaci ed efficienti. Papa Francesco ha detto che non devono esserci poveri e non c'è peggior povertà di quella che non ci permette di guadagnarci il pane, che ci priva della dignità del lavoro. Con questa straordinaria manovra (perché è straordinaria) noi non regaliamo alcuna illusione; noi offriamo un'opportunità ai dimenticati, a chi non è raccomandato, a coloro che vogliono vivere - e hanno il diritto di farlo - dignitosamente, perché nessuno deve restare indietro. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Catalfo. Signor Presidente, cercherò di riassumere e di rispondere agli interventi dei senatori che mi hanno preceduto. decreto-legge in discussione è un'ondata demagogica, che il nostro provvedimento è confuso, che gli altri Paesi non lo hanno messo in atto come stiamo facendo noi, che non prevede controlli efficienti

un provvedimento legato al contesto elettorale e la dimostrazione è che il MoVimento 5 Stelle sin dall'inizio, quindi dal primo ingresso

il reddito di cittadinanza. Non solo lo ha proposto, ma lo ha portato avanti per cinque anni malgrado fosse all'opposizione. È chiaro che il primo punto del programma alle elezioni politiche del 2013 2013 e del 2018 diventa uno dei primi punti da portare avanti con urgenza per questa maggioranza e per questo Governo.

di famiglie e bambini in povertà; una povertà che è aumentata nel corso degli anni che quindi le politiche messe in atto dai precedenti Governi non sono riuscite a contrastare: una povertà che certamente influisce non solo sulla vita

un provvedimento necessario e urgente. Mi è stato contestato il fatto di averlo definito un provvedimento storico. È un provvedimento storico, in primo luogo perché l'attuazione degli articoli della Costituzione italiana; in secondo luogo, perché contrasta la povertà che purtroppo affligge il nostro Paese; in terzo luogo, perché fa il primo importante investimento, dopo decenni, nelle politiche attive del lavoro e nei centri per l'impiego.

i centri per l'impiego aumentando il personale con ben 7.600 addetti; aumentiamo le risorse strutturali; implementiamo le piattaforme informatiche, quindi consentiamo l'interoperabilità delle banche dati, e questo è un altro importantissimo investimento che non si era fatto in Italia negli ultimi anni.

mettiamo in rete tutti quegli attori che, a vario titolo, si occupano in Italia di erogazione di servizi per l'impiego, quindi anche le agenzie per il lavoro private, che hanno un ruolo all'interno dell'erogazione dei servizi per i beneficiari di reddito. Ampliamo, tra l'altro, i servizi a tutti coloro i quali - i cosiddetti *working poor* - si trovano in una situazione di occupazione, ma in un

È stato detto in quest'Aula che questa riforma è difforme da quanto realizzato negli altri Paesi europei. ha effettuato un'indagine conoscitiva importante sul contesto nazionale ed europeo dei servizi per l'impiego e si è recata, a tale scopo, in visita in Germania e in Francia per vedere come gli altri Paesi hanno strutturato l'inserimento lavorativo e i centri per l'impiego. In Germania, ad esempio, dove la situazione era simile a quella italiana, hanno collegato i servizi sociali dei Comuni e i centri per l'impiego in un unico ufficio chiamato *job center*, che prende in carico il cittadino

aiuto fornito dai servizi sociali dei Comuni, ma è anche vero, dall'altra parte, che la persona si deve rendere proattiva e capace di poter poi avere una vita indipendente e quindi di essere inserita nel contesto lavorativo. Per tale motivo, noi colleghiamo i servizi sociali dei Comuni ai centri per l'impiego e creiamo anche una rete, che è stata ancor più

anche incrociata, del soggetto. Detto questo - e rispondo anche ad alcune osservazioni del Gruppo del Partito Democratico - non si può lasciare

non sia efficace ai fini dell'inserimento nel contesto sociale lavorativo e della futura vita indipendente del beneficiario (indipendente nel senso che può avere un lavoro e un salario futuro).

che fece un rapporto. Se dunque si va a leggere attentamente tale rapporto, si comprende che la difficoltà dell'inserimento della presa in carico non efficace e non efficiente da parte dei servizi sociali. È chiaro, quindi, che va fatto un collegamento tra la prima presa in carico e l'aiuto all'inserimento lavorativo, necessario per avere poi un effetto e un impatto positivo sul cittadino e sul beneficiario che viene accompagnato.

nei servizi per l'impiego, nelle prese in carico e nel reale, effettivo ed efficace aiuto all'inserimento lavorativo.

con cui gettiamo le basi per un nuovo Stato sociale, realizzando un nuovo statuto delle garanzie e non solo del lavoro, basato sul fatto stesso di essere cittadini. un concetto idoneo a ridisegnare il diritto all'esistenza e a garantire una piena autodeterminazione dei cittadini. *(Applausi

come spesso viene sottolineato dalle opposizioni - è stato fatto anche oggi - la Lega e il MoVimento 5 Stelle sono due partiti che su molte questioni e su molti argomenti hanno sensibilità diverse,

Molto spesso - è stato fatto anche oggi - ho sentito criticare la Lega e il Governo, tacciati più volte di considerare lo straniero un furbo a prescindere.

tant'è che in prima lettura al Senato è stato approvato un emendamento che prevede che il cambio di residenza venga certificato da un apposito verbale della polizia locale in caso di separazione o divorzio avvenuto successivamente al 1° settembre 2018. Questo emendamento si è reso necessario proprio le numerose segnalazioni giunte dai sindaci, che hanno evidenziato come il numero dei cambi di residenza fosse cresciuto in maniera esponenziale. Questi cambi di residenza - lo sottolineo - erano richiesti sia da italiani che da stranieri. È stato approvato anche un altro emendamento, che ha provocato forse qualche mal di pancia in più alle opposizioni. Mi riferisco a quello relativo alla presentazione della certificazione delle proprietà immobiliari del Paese d'origine da parte dei cittadini UE. Vorrei soffermarmi nuovamente su questo punto, anche se l'avevo fatto in prima lettura in sede di replica, perché tanti non hanno capito il senso. La richiesta della certificazione si è resa necessaria per una questione di equità nei confronti degli italiani e non perché si considera lo straniero un furbo a prescindere, come è stato detto più volte. Mentre per beneficiare dei servizi sociali dei Comuni l'italiano è soggetto al controllo puntuale e immediato al catasto dei beni immobiliari di proprietà e senza alcun costo in capo all'ente, ciò non avviene per lo straniero extra UE che, grazie ai Governi di sinistra, se l'è sempre cavata con una semplice autocertificazione. Il fatto è che per mancanza di strumenti o per la carenza di risorse finanziarie i Comuni non sono in grado di fare gli opportuni controlli sulla veridicità delle informazioni fornite.

va incontro anche alle critiche mosse più volte dall'opposizione legate all'appesantimento delle incombenze in capo ai Comuni e l'applicazione del criterio è già stato sperimentato con esiti positivi in molti Comuni dove la Lega governa. Non ci si ferma qui perché tante altre sono le migliorie inserite. Ad esempio, rispetto al testo base, che prevedeva per i lavori socialmente utili solamente otto ore settimanali, siamo passati da un minimo di otto a un massimo di sedici ore, previo accordo consensuale tra le parti. Queste e tante altre modifiche hanno portato a migliorare il decreto-legge con la finalità di andare incontro a richieste e osservazioni pervenute anche dalle stesse opposizioni. Veniamo a quota 100. Ne parlo con infinito orgoglio perché è l'ennesima promessa agli italiani che aspettavano da anni una risposta concreta. Mi perdoni l'opposizione, ma non accettiamo lezioni da chi ha votato e sostenuto la legge Fornero, compresa Forza Italia, da cui sono arrivate le critiche più pesanti. *(Applausi 100 non è una finestra per pochi, ma un finestrone che in tre anni consentirà a quasi un milione di persone di andare in pensione a un'età accettabile, un'età che consentirà loro di dedicarsi alle famiglie e ai nipoti. La figura dei nonni e della famiglia è, ancora una volta, al centro della nostra azione politica. Di questo siamo fieri e ne andiamo orgogliosissimi. Quota 100 è stata una scelta consapevole per cominciare a svuotare il bacino della legge Fornero e dare respiro al mercato del lavoro. Il numero di richieste di adesioni ci dà una sola risposta: che abbiamo ragione. A chi critica parlandoci di quota 41, rispondo che il sistema economico e lavorativo non avrebbe retto se, in base ai dati, avessero chiesto di andare in pensione tutte insieme le 700.000 persone che ne avrebbero avuto diritto. diritto. Non dimentichiamo inoltre - e l'abbiamo attuato - il blocco dell'aumento dell'aspettativa di vita per le pensioni anticipate. Di questo ne beneficeranno tutti. Vogliamo parlare anche della questione dei dipendenti pubblici, che molto spesso è stata sollevata sia in Commissione che in Aula.

linea con il disegno di legge concretezza, che è stato tanto criticato, ma che prevede assunzioni mirate, rivolte proprio ai giovani con specifici requisiti, volte a migliorare ed efficientare la macchina amministrativa pubblica. Inoltre, da novembre ci sarà lo sblocco del *turnover*, con il rapporto tra coloro che vanno in pensione e i nuovi assunti pari a uno a uno, e i posti di lavoro che verranno liberati grazie allo sblocco delle assunzioni - sempre ad opera di questo Governo - consentiranno a tanti giovani di entrare nel mondo del lavoro.

in tre anni ci saranno un milione di vincitori che si meritano questo premio; persone che sono rimaste in attesa per anni per colpa della legge Fornero. E poi vorrei dire basta: basta con la continua accusa che la Lega campa di meri *spot* elettorali. Ormai non siete neanche più credibili, e sapete perché? Perché sono i numeri che parlano da soli. Il 26 febbraio, durante la mia replica in prima lettura, avevo dato un numero: 67.738, ovvero il numero delle richieste presentate per quota 100. Oggi, a distanza di un mese, queste richieste hanno raggiunto quota 103.000: circa 35.300 richieste in più in un solo mese. Gli italiani sanno benissimo che quota 100 non è uno *spot* ma un'ulteriore promessa promessa mantenuta e a darci ragione sono i quasi 36.300 lavoratori dipendenti che hanno fatto richiesta per quota 100; i 35.800 dipendenti pubblici che hanno fatto richiesta; gli 8.500 commercianti e i quasi 9.000 artigiani. Va sottolineato inoltre che quota 100 è una facoltà, non un obbligo, e i 103.000 italiani che hanno fatto richiesta lo hanno fatto liberamente, senza alcuna costrizione. Concludo, Presidente, sostenendo convintamente che quota 100 è un ulteriore esempio di come la Lega sia passata dalle parole ai fatti: l'ennesima promessa mantenuta, e ancora una volta le percentuali ci danno ragione. Onorevoli colleghi, la Presidenza, analogamente a quanto già stabilito in sede referente, dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 1.5, 2.3, 2.4, 2.40, 3.4, 4.6, 4.10, 6.1, 6.50 (già 7-*ter*.l), 6.2, 6.3, 7*-ter*.0.1, 7*-ter*.0.2, 8.1, 10.5,

in quanto non correlati alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, Forza Italia è stata sempre attenta alle fasce più deboli della popolazione. Lo abbiamo sempre dimostrato nei fatti, lo sosteniamo e ne abbiamo dato prova anche con questo provvedimento perché tanti e tanti sono stati i nostri emendamenti

nel futuro. Purtroppo il provvedimento non porterà nemmeno alla diminuzione della disoccupazione e tutte le strutture che dovrebbero essere messe in condizione di prendersi in carico i beneficiari del reddito di cittadinanza, come ha già detto chiaramente la senatrice Catalfo, non sono pronte. Ciò dimostra ancora una volta che il provvedimento servirà soltanto

ci dispiace che gli amici della Lega applaudano contro Forza Italia, perché noi in realtà ci eravamo presi un impegno, firmato da noi e dagli amici della Lega,

non prenderà l'intero importo, ma vedrà riconosciuta la pensione rispetto agli anni di versamento dei contributi con riferimento alla legge Fornero. Si tratta quindi di un'ennesima finestra e questo accade perché è una misura *spot* che, come tutte le altre misure del Governo, che vedono due forze politiche in contrasto tra loro, si è dovuto procedere con la regola del ribasso. Noi invece avremmo voluto farlo in maniera efficace affinché tutti andassero in pensione e non soltanto il signor Walter. Per carità, siamo

che includeranno ed escluderanno, ma non aumenteranno i diritti. Il tema dei diritti è molto importante in uno Stato democratico e queste norme non supereranno la legge Fornero.

non costruite una norma che va ai diritti sociali, tant'è che i suoi beneficiari non vi andranno tutti.

quindi per tutti. Chiudo dicendo che è molto facile - lo sarebbe per tutti i Governi - fare norme che includono ed escludono altre persone. Faccio un solo esempio, riprendendo il tema della disabilità: perché non si è messo mano a una scala di equivalenza che dia di più alle famiglie che hanno persone con disabilità?

Il rappresentante del Governo non intende intervenire

Grazie Presidente. ultimo periodo, di sostituire le parole: «di età inferiore al predetto requisito anagrafico» con le seguenti: «a prescindere dall'età anagrafica della persona in condizione di disabilità

A fine mese questi lavoratori riusciranno a interloquire e ringraziare il vice *premier* Di Maio? Sono sfruttati, o no? Qual Qual è la vittima e qual è il carnefice nel nostro Paese? È lo Stato, o sono solo le imprese private? Come è possibile, dopo l'adozione del

vero o falso. Se è vero, mi aspetto che il ministro Di Maio chieda scusa non a me, ma a quei lavoratori, e che voi del MoVimento MoVimento 5 Stelle riandiate in tutte le piazze del Paese a chiedere scusa per quanto sciacallaggio avete fatto, finalizzato all'organizzazione del consenso. Vergognatevi, avete bisogno di dignità politica.

Presidente, inizio con l'illustrare gli 2.10, 2.11 e 2.12, con i quali il Gruppo Fratelli d'Italia chiede di escludere dal reddito di cittadinanza le persone condannate per peculato, concussione e corruzione. Spetta a voi, adesso, la responsabilità di decidere.

Grazie a migliorare un testo che ci vede palesemente contrari, perché si tratta soltanto di un provvedimento di bandiera, un provvedimento che unisce le due bandiere dei due partiti al Governo facendone, di fatto, due mezze bandierine che non porteranno a niente. Quello che ci dispiace molto e che ci era stato garantito durante la discussione in Commissione lavoro è che sui temi della disabilità e del sostegno alle famiglie numerose

12 milioni di euro. Avete spostato, su 7 miliardi di investimento per le politiche di contrasto alla povertà, 12 milioni di euro (praticamente una minuzia) sulle famiglie. Allora vi dico: basta parlare di famiglie, di politica per la famiglia e di sostegno alle famiglie. Proviamo a fare cose concrete. Questo poteva essere un provvedimento che lasciava un segnale importante per le famiglie più povere del Paese. Non l'avete fatto e state sbagliando clamorosamente. *(Applausi dal Gruppo

dalle repliche del Governo, per quale motivo vi siete così intestarditi nel voler chiudere o sbattere addirittura la porta in faccia alla disabilità.

punto. Colleghi, alla Camera la maggioranza, dopo aver visto che in fila per conseguire il reddito di cittadinanza c'erano anche noti delinquenti, ha introdotto una norma secondo la quale tra i requisiti per ottenere tale reddito ci deve essere anche la mancata sottoposizione a misura cautelare personale. Va bene, ma c'è un piccolo problema, come ho detto anche in discussione generale: intanto non è detto che tutti debbano per forza essere sottoposti a misura cautelare

In dottrina si fa l'esempio, piuttosto concreto, del marito uxoricida che uccide la moglie perché è geloso, perché la scopre in flagranza che confessa e si costituisce. A quel punto non c'è pericolo che ripeta il reato perché la moglie non c'è più; non c'è pericolo che scappi perché si è costituito; non c'è pericolo che inquini le prove perché ha confessato; non è sottoposto neanche un giorno a custodia

si chiede di escludere dal beneficio chi ha subìto una condanna per delitti non colposi a una pena non inferiore a due anni, e ancora meglio il 2.9, si dice che i due anni possono essere anche il frutto delle somme delle condanne perseguite. Facciamo - ad esempio - l'ipotesi di chi vive

spero che quest'Assemblea si renda conto di ciò che stiamo votando ed esprima un parere favorevole su almeno uno di questi due emendamenti.

in Senato, abbiamo ribadito e ribadiamo nuovamente. Davanti al silenzio del sottosegretario Cominardi e del Governo rispetto al quesito che abbiamo posto e che ha posto anche

cosa intendono fare sul serio, e non con dichiarazioni altisonanti, con le famiglie che hanno figli disabili e con le famiglie numerose con minori. Ripeto che attendiamo una risposta e speriamo di averla presto.

reati, in modo da poter mettere il Senato nelle condizioni di decidere se c'erano alcuni specifici reati per cui escludere le persone dall'accesso al reddito di cittadinanza. Mi riferisco a reati particolarmente odiosi come la pedofilia, l'omicidio, l'infanticidio, la mutilazione degli organi genitali, la riduzione in schiavitù, la prostituzione, lo sfruttamento dei minori, l'accattonaggio, il sequestro di persona, la violenza sessuale, la corruzione, la rapina, il sequestro. Noi chiedevamo al Senato di esprimersi rispetto alla nostra richiesta di escludere questi odiosi reati dalla possibilità di accedere al reddito di cittadinanza *(Applausi dal Gruppo possibilità, ma rimanga agli atti che era la nostra richiesta e la responsabilità è in capo a chi ha votato contro i nostri emendamenti. Senatore Ciriani, vorrei solo farle presente che gli emendamenti cui lei fa riferimento non sono stati dichiarati inammissibili, ma sono rimasti preclusi dalla reiezione di un emendamento precedente. Dico questo solo

un'eventuale cifra che avrebbe dovuto incidere all'interno del contesto del provvedimento veramente per pochissimi milioni, ma avremmo dato un segno di particolare attenzione verso le famiglie in difficoltà per la presenza di un disabile. Mi auguro ancora che ci possa essere un ravvedimento, ma non credo che ci sarà.

alla maggioranza e al Governo che in questo emendamento si propone l'approccio che noi abbiamo cercato di proporre - scusate il gioco di parole

ma mette a disposizione una banca dati presente su tutto il territorio nazionale che raccoglie offerte di lavoro.

Mi vergognerei a parlare di basse retribuzioni, fossi in lui, visto che continua a pagare le persone 4 o 3,50 euro l'ora. Non è una questione di mercato

esisteva già la schiavitù nella Virginia del 1800 e si poteva avere un campo di cotone pieno di lavoratori che non si pagavano, ma io non l'avrei fatto, perché è una questione etica, anche se la legge lo permette.

mi sento coinvolto e intervengo con una certa determinazione per aver svolto la funzione di sindaco per dieci anni. Anche con questo provvedimento, così come in altri, si prevedono maggiori carichi di lavoro per le verifiche, i controlli e tutti gli accertamenti della residenza, cui è tenuto il Comune, senza dare alcun contributo. ridotti i trasferimenti ai Comuni e adesso si aumentano gli oneri per gli stessi. Ritengo che ciò sia veramente poco dignitoso e poco rispettoso da parte del Governo nei confronti delle autonomie locali. Sono certo che anche questa volta l'emendamento

invito il Ministro, che conosce la situazione del Sud e non solo, con riferimento alle difficoltà delle casse dei Comuni, a voler provvedere in un atto separato e successivo, date le tante occasioni che ci saranno per l'applicazione di questo

frase: «comprensiva dello stato di attuazione delle singole misure e dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1.» L'articolo 10 si concentra sul monitoraggio. Noi crediamo

misura di questa portata, si abbia bisogno di una verifica e di una sorta di vera clausola valutativa, che può essere esercitata solo ed esclusivamente da un organo terzo; terzo; altrimenti il monitoraggio fatto dal Ministero altro non è che una sorta di autocertificazione. Noi non chiediamo questa terzietà per per il dibattito politico, per avere vantaggi da un punto di vista politico e poter dire che avevamo ragione o che ve l'avevamo detto. In una qualsiasi impresa, attività privata o pubblica, per un qualsiasi provvedimento normativo è necessario e dispensabile capire se quelle finalità vanno a impattare così come sono state previste. Se, invece, impattano in un modo diverso e discordante rispetto alle finalità, si può intervenire. Questi sono i motivi e i presupposti per cui abbiamo suggerito in prima lettura, in seconda lettura alla Camera, e in terza lettura ancora adesso, di creare uno spazio all'interno dell'articolo 10 per dare la possibilità a esperti o tecnici di migliorare il vostro provvedimento. Questo, purtroppo, non è stato attuabile e nei prossimi mesi non sapremo effettivamente dove andare a migliorare e che cosa rettificare nel più breve tempo possibile per evitare tutta una serie di storture. Anche nel caso specifico, non riusciamo a capire perché vi intestardite in questo modo. Una risposta poi ce la diamo: perché siamo alla sagra della autocertificazione.

all'articolo 10 e riguarda i monitoraggi, nel dettaglio entra nel merito dei monitoraggi rispetto alle famiglie con persone con disabilità e soprattutto di famiglie che hanno al loro interno la figura del *caregiver* familiare, cioè di quella persona che si prende cura

del *caregiver* familiare sono *in itinere* all'interno della Commissione, sono allo studio. Quindi, approvando un emendamento del genere, al di là della dimostrazione dell'attenzione, che - ribadisco - pare comunque continuare a non esserci nei confronti delle famiglie con disabili e soprattutto della figura del *caregiver*, che come lavoratore deve avere necessità di un'attenzione particolare,

propositiva da parte delle opposizioni, che in questo caso non fanno opposizione, appunto, ma fanno proposizione costruttiva.

destinato altri 25 milioni di euro, nell'arco di tre anni, ad ANPAL per spese di funzionamento non ben definite, in barba ai princìpi di trasparenza anche del Governo stesso. Qualche giornale ha fatto un po' di illazioni

Il personale precario negli ultimi anni ha partecipato anche a procedure di selezione ad evidenza pubblica secondo le decisioni dell'azienda, sottoponendosi a prove selettive, a volte per la stessa posizione ricoperta in precedenza.

anche noi continueremo a stare al fianco del personale di ANPAL Servizi S.p.A. dei sindacati che hanno seguito il percorso di stabilizzazione nel 2017, e del coordinamento dei precari: tutte persone che meritano in questa fase l'assunzione.

senatrice Malpezzi

che gli insegnanti vogliono andare in pensione e immaginiamo proprio che le domande di pensionamento saranno tantissime. Il problema - e mi rivolgo al Governo - è che non avete pensato chi metterete in classe, perché non avete attuato alcun sistema che garantisca che, a fronte di un numero tanto elevato di insegnanti che andranno in pensione, ce ne siano altri pronti a garantire la continuità didattica e non avete dato diversi ordini di risposte. Che cosa farete con gli insegnanti che hanno più di trentasei

protestando, perché, a fronte di cattedre scoperte, non ci sarà un sistema pronto a reinserire altri docenti all'interno del mondo del lavoro. Ancora, vi abbiamo dato un altro suggerimento: fate in in modo di far fare i cosiddetti passaggi di cattedra ad insegnanti abilitati, che hanno già vinto il concorso e possono andare ad insegnare in altri ordini di scuola. Liberereste posti e avreste già personale

per garantire la continuità didattica. L'avete abolito: è una scelta politica, ne abbiamo già discusso tante volte. Il problema è che non avete messo nulla in sostituzione, per cui a settembre la nostra scuola sarà un disastro e sarà solo ed esclusivamente colpa vostra.

su quota 100 rispetto al mese scorso possiamo oggi fare qualche riflessione, partendo dai numeri delle domande. Appare evidente che questa misura produrrà effetti molto limitati sul fronte del ricambio generazionale nel mondo del lavoro. Importanti studi ci dicono che nel privato ci sarà un ricambio di uno a dieci e questo per la semplice ragione che a chiedere la pensione sono dipendenti di aziende in difficoltà e che lo saranno ancora di più per la recessione economica. Sulle domande presentate dagli autonomi, il rischio molto concreto è che continueranno a svolgere la loro mansione lavorativa, intestando l'attività a familiari. Nella pubblica amministrazione in molti hanno denunciato i problemi che avranno il mondo della scuola e la sanità. Qui, anche con tutta la buona volontà, per avere un ricambio ci vorranno anni, quelli necessari per bandire e realizzare i concorsi pubblici, per procedere poi con le assunzioni. Vi è poi il tema dello squilibrio di genere: 75.000 domande maschili contro appena 25.000 femminili. Questo perché con quota 100 non è stato affrontato il problema delle donne che hanno meno contributi e a cui non viene riconosciuto il lavoro di cura e accudimento familiare. Soprattutto, ciò avviene nella cornice di una nuova recessione economica. Se l'obiettivo era creare nuovo lavoro, forse non era meglio destinare queste risorse per il taglio del cuneo fiscale o sotto forma di agevolazioni per le imprese? Permane infatti il grande problema della sostenibilità del sistema pensionistico. Il punto vero è che in Italia si parla di pensioni sempre dal punto di vista di chi ci vuole andare e mai da quello di chi quelle pensioni dovrà poi pagare. Sul reddito di cittadinanza, come abbiamo già detto in prima lettura, siamo favorevoli a misure di contrasto alla povertà, simili a quelle di tanti altri Paesi europei. Tuttavia, abbiamo forti perplessità sul come è stata costruita la misura. La prima riguarda il collegamento tra povertà e lavoro. La povertà è un concetto molto più vasto e complesso. La povertà è quella, ad esempio, di una madre *single*, con figli piccoli, in assenza di strutture e servizi pubblici adeguati. È la condizione di marginalità sociale in cui versano minori che non hanno occasioni e strumenti di apprendimento e che sono a rischio dispersione scolastica. C'era quindi bisogno di uno strumento che affrontasse il problema coinvolgendo i servizi sociali dei Comuni e non scaricando tutto sui centri per l'impiego, che non hanno il personale e la formazione adeguata per farsene adeguatamente carico e che non funzioneranno neanche per la ricerca di lavoro. Mancano le strutture adeguate, il personale, i computer e anche i nuovi *navigator* non porteranno valore aggiunto, visto che è diventato semplice personale di supporto tecnico. Dai dati sul reddito quello che più colpisce è l'assenza dei giovani. Pochissime domande, gli *under* 30 sono solo il 6,8 per cento, eppure il reddito è sempre stato raccontato come lo strumento per mettere in moto una generazione. Non sta succedendo e non succederà. Per incoraggiarli ad andar via di casa, a cercare la strada dell'indipendenza, la legge andava scritta in altro modo. La verità è che ci voleva tempo per coinvolgere le parti sociali, per non sovrapporre povertà e lavoro, per riformare i centri per l'impiego, per bandire concorsi pubblici per i *navigator*, per avere controlli e verifiche efficaci sui percettori del reddito. Per questi motivi di merito del provvedimento, dovremmo votare contro. Tuttavia, diamo atto al Governo di aver accolto la clausola di salvaguardia che consentirà ai cittadini delle Province autonome di poter optare tra il percorso nazionale e il reddito d'inclusione provinciale, che noi valutiamo molto più efficace e rispondente alle necessità dei cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà o di fragilità sociale. Esprimeremo pertanto un voto d'astensione. noi ci asterremo su questo provvedimento: è la sintesi di un giudizio che abbiamo già espresso in prima lettura e che abbiamo ribadito nel passaggio alla Camera. Per noi l'astensione vuol dire, innanzitutto, non contrarietà rispetto ad uno strumento che, nella sua ispirazione di fondo, ha un obiettivo ambizioso che è quello di contrastare le povertà e di immaginare una misura di sostegno al reddito. Per noi ogni euro del bilancio pubblico che viene messo a disposizione per fare questa operazione è un euro ben speso, soprattutto in un Paese nel quale le povertà sono aumentate. Lo si dice spesso con molta facilità e persino con un pizzico di retorica, ma è la fotografia reale del Paese. Ce lo dicono le statistiche ma dietro quei numeri, così freddi, si nasconde la vita reale delle persone. Stiamo parlando della povertà assoluta, di coloro che non arrivano alla fine del mese (molte di queste famiglie non arrivavo neanche alla terza settimana). Stiamo parlando, caso con una categoria un po' algida propria degli istituti di statistica, della cosiddetta povertà relativa il che vuol dire sostanzialmente quella condizione nella quale le persone non possono fare quelle cose che magari altri hanno la possibilità di fare e nel non farle stanno compromettendo la propria dignità. Sono persone che non possono possono svolgere una vita normale, non possono assicurare a sé stessi, ai propri cari e ai propri figli delle condizioni dignitose di vita. Molto spesso, anche genitori che non riescono neanche a fare la festa di compleanno per i propri bambini e quando in un Paese che si bea,

e cercare di rimpicciolire quelle faglie che si sono allargate in ragione della crisi economica e sociale molto pesante degli ultimi dieci anni;

generazioni. Questa è la ragione per cui noi sentiamo di guardare con interesse a questo provvedimento e lo abbiamo fatto sin dall'inizio. I miei colleghi sanno che in Commissione lavoro lo spirito con cui abbiamo proposto e affrontato la fase emendativa è stata esattamente questa, cioè quella di non contrastare in modo pregiudiziale, ma di capire come modificare in senso positivo un provvedimento che avesse innanzitutto questo tipo di principio e di ambizione, che ci sentiamo di condividere. Aggiungo anche - l'ho già detto in precedenti interventi, ma mi sento di ribadirlo che ci sentiamo molto lontani da quelli che propongono la tesi del divano, cioè da quelli che dicono che il reddito di cittadinanza favorirebbe il poltrire dei nostri giovani sul divano, perché disincentiva la ricerca di un lavoro in quanto l'integrazione al reddito è molto vicina al livello medio dei salari. Questa è una tesi non solo un po' curiosa, ma persino offensiva, perché vuol dire che chi la propone non conosce la condizione di molti giovani e anche di molti meno giovani di questo Paese, ma soprattutto perché non mette al centro un altro tema: se il livello del reddito di cittadinanza è molto vicino ai salari medi del Paese, vuol dire che l'Italia ha una gigantesca questione salariale da risolvere e che bisogna aumentare M5S)*. Credo che sia questo il centro della discussione che dobbiamo fare. Detto questo, visto che dall'opposizione ci prendiamo la libertà e - fatemi dire - persino l'autonomia intellettuale e politica di astenerci di fronte al provvedimento simbolo di un Governo che noi contrastiamo, con la stessa libertà ci sentiamo di dire - l'abbiamo già detto nei passaggi precedenti - quali sono gli enormi buchi e le contraddizioni del provvedimento, che, per una strana eterogenesi dei fini, rischiano di portarlo in una direzione diversa, se non in alcuni casi opposta agli obiettivi che il legislatore si prefigge e quindi che la maggioranza si è posta.

rischia di tenere fuori i senza fissa dimora, cioè gli ultimi degli ultimi della nostra società? Perché non è stato messo sufficientemente al centro il tema dei minori poveri? Perché non avete fatto uno sforzo adeguato (anche se qualche piccolo ritocco lo avete fatto) rispetto a una grande questione, cioè al fatto che molte famiglie, avendo al loro interno e nel loro nucleo persone disabili, assommano a una condizione materiale molto pesante, che fa diventare persino più drammatica la loro condizione di povertà, anche una condizione non squisitamente materiale, cioè una condizione umana? Perché non avete

numericamente a trazione MoVimento 5 Stelle, ma politicamente guidato ormai dai colleghi della Lega, è evidente che questo criterio è stato

ha a che fare con persone migranti che vivono regolarmente nelle nostre città e nelle nostre comunità. e nelle nostre comunità. C'è poi tutto il tema della gestione dello strumento, di questo meccanismo per cui si creeranno precari a mezzo di precari; l'idea che non abbiate risolto la questione dei precari dell'ANPAL a noi sembra un'assurdità e una contraddizione. Il provvedimento che dovrebbe far emergere dalla condizione di frammentazione del lavoro e di precarietà dovrebbe essere gestito da chi continua a restare precario e rispetto al quale non è stata trovata una soluzione di stabilizzazione.

Questa non è una quota 100, è soltanto un passaggio sperimentale e soprattutto non risolve i nodi strutturali del sistema pensionistico, che riguardano le carriere discontinue delle donne e dei giovani, e non risolve il problema dei lavori usuranti, oltre al fatto che non avete messo mano alla questione degli esodati. Per queste ragioni noi ci asterremo. Ci sono luci, noi le vediamo, ma ci sono molte ombre. Ci auguriamo che il Governo - questa è la richiesta che facciamo - possa in qualche modo risolvere i tanti problemi rimasti aperti nella fase di implementazione e di attuazione del decreto-legge.

non riusciva a mettersi d'accordo per quanto riguardava gli emendamenti presentati. Ciò era abbastanza evidente, dato il numero degli emendamenti presentati al reddito di cittadinanza da parte della Lega e gli emendamenti su quota 100 da parte del MoVimento 5 Stelle. Quando finalmente, dopo una riunione a Palazzo Chigi, siamo riusciti a tornare in Commissione e a iniziare la discussione, ma soprattutto a illustrare gli emendamenti, partito da questo ramo del Parlamento, pensavamo che ci si potesse lavorare; pensavamo soprattutto di poter dare il nostro contributo. in pochissimo tempo abbiamo invece capito, perché ci è stato spiegato, che tutto sarebbe stato rivisto e corretto alla Camera, perché erano ancora in corso trattative all'interno della maggioranza e al tavolo con le Regioni. quindi impossibile contribuire. Abbiamo guardato con fiducia i lavori svolti alla Camera ma alla fine abbiamo dovuto constatare, per l'ennesima volta, l'ulteriore presa in giro. Vi avevamo con forza sottolineato

nei confronti delle persone disabili, per non parlare, poi, delle famiglie numerose. So che dà particolarmente fastidio al Movimento 5 Stelle, ma di fatto questo è un provvedimento assistenziale

e gli interventi sociali: sono due interventi completamente diversi, che non possono stare insieme. Soprattutto,

Nella zona del padovano la CGIL dice che li dovranno restituire, mentre la CISL dice di no; questo in base a una circolare che è stata inviata dall'INPS, che evidentemente non ha chiarito

Ma come pensate che i Comuni possono reggere all'ondata che ci sarà? Ve l'ho detto anche nella fase della prima lettura: la presa in carico è una cosa importante che viene fatta dai servizi sociali, e spesso e volentieri non si riduce alla singola persona, ma è una presa in carico anche del nucleo familiare. Non avete poi dato disposizioni per quanto riguarda l'aumento del personale che dovrà occuparsi di queste cose. Avete negato qualsiasi tipo di modifica per gli incentivi alle aziende che andranno ad assumere le persone con reddito di cittadinanza, tra l'altro una contraddizione, perché l'azienda che dovesse assumere una persona che prende il reddito di cittadinanza probabilmente selezionerà quelli che il reddito di cittadinanza hanno appena iniziato a prenderlo,

Abbiamo poi cercato più volte di dirvi anche che dovevano essere incrementati i contributi per chi decidesse di intraprendere la strada dell'autoimpresa, perché crediamo che

sottolineare particolarmente che questa mattina, durante la discussione generale, ho sentito parlare di poveri quasi con voce

porta a capire che qui non c'è un ragionamento sulla povertà. Le associazioni che sono venute in Commissione a parlarci

per noi - mi spiace dirlo - è stato un mese perso nel provare a suggerire e a indicare modifiche migliorative e ragionevoli ad un decreto-legge nato male, sin dall'inizio. Siamo stati presi in giro. Il ministro Di Maio in queste settimane ha auspicato un confronto, un ascolto attento, possibili convergenze sulle politiche sociali e sulle politiche del lavoro: è una grande bugia, una grandiosa preso in giro. I confronti si fanno alla luce del sole, si fanno qui in Aula e soprattutto nelle Commissioni e non certo ricorrendo al decreto-legge. in esame avete fatto dichiarazione altisonanti. Avete parlato di cancellazione della povertà, quando oggi la crisi economica incombe sul Paese: lo ha certificato solo ieri pomeriggio il Fondo monetario internazionale. Siamo in recessione senza che abbiate mosso un dito. I poveri non scompariranno - ahimè per le famiglie - ma rischieranno di aumentare nei prossimi mesi. Avete parlato di riforma strutturale del *welfare* e anche questa mattina ho ascoltato questo passaggio. In realtà, avete introdotto un provvedimento con risorse a debito; avete introdotto un principio costituzionale un po'

Non avete poi riformato il *welfare* ed il provvedimento si poggia su infrastrutture storicamente fragili, *in primis* i centri per l'impiego, che sono quelli che conosciamo. Avevate annunciato una riforma strutturale; l'aveva annunciato lo stesso Di Maio. Abbiamo avviato una serie di audizioni in Commissione, non ancora concluse e di cui non si conosce lo sbocco: una proposta di legge o una riforma contenuta nel decretone? Se la riforma annunciata dal ministro Di Maio sui centri dell'impiego fosse questa, davvero potremmo dire di essere a «Scherzi a parte». Avete fondato il provvedimento sulle piattaforme digitali, ma è noto come sia difficile per le persone più fragili accedere a queste ultime. Sappiamo anche - lo dicono anche gli esperti - che quel potenziamento delle piattaforme digitali cui auspicate nel decreto richiederà anni di tempo. Avete azzerato il lessico, le parole chiave che hanno percorso in questi anni il dibattito pubblico e scientifico a livello europeo. Neppure avete fatto proprio il linguaggio e il lessico del pilastro europeo dei diritti sociali: *welfare* di comunità, prossimità, multidimensionalità, ascolto, presa in carico, responsabilità, reciprocità, parole escluse dal dibattito e neppure presenti nel decreto.

è da lì che occorreva ripartire perché, quando si parla di *welfare* più giusto e più inclusivo e di attenzione alle fragilità, parliamo di territori. Sono le comunità che che si prendono carico delle fragilità; sono le reti di comunità, le reti di terzo settore, i nostri amministratori e i nostri assessori che voi avete trascurato. In questo provvedimento chiedete impegni agli enti locali senza offrire alcunché, senza offrire risorse e senza aiutarli in un processo di nuova infrastrutturazione. Avete dimenticato la sussidiarietà orizzontale (mi stupisco dei colleghi della Lega, che sulla sussidiarietà nei decenni scorsi hanno fatto grandi battaglie anche ideologiche) le realtà civili e religiose. Non avete neppure accennato alla necessità di riconquistare una cultura di progettazione condivisa a livello locale, uno strumento prezioso per contrastare la povertà, per ridurre la frammentazione della comunità; sono parole care a noi tutti, a coloro che hanno a cuore il *welfare*, la povertà e le fragilità; come anche coprogettazione, reti, comunità, presa in carico, collaborazioni, sinergie persino con le imprese (chiamate invece in un gioco strano e artefatto). Avete dimenticato persino la sussidiarietà verticale, scavalcando le Regioni e i Comuni, recuperati malamente in "zona Cesarini". Non pensiamo sia un caso; non credo che tutto questo sia un caso il decreto sia dovuto a qualche distrazione. I vostri provvedimenti si nutrono del pregiudizio e del sospetto sul quale avete costruito un'impalcatura antropologica - vedi i vari decreti concretezza eccetera - fondata sulla diffidenza, sul cittadino da solo, una monade, disperso, senza comunità e senza reti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Un cittadino da solo che guarda il suo *leader* in attesa della soluzione finale. Nondimeno avete introdotto una normativa punitiva verso i poveri che lascia sconcertati. Avete persino introdotto il controllo sui consumi. Sapete bene che i cosiddetti furbetti si contrastano con i controlli che - ahimè - non saranno incrementati con la soluzione di una piccola pattuglia, generosa e coraggiosa, di carabinieri e finanzieri. I controlli si incrementano assumendo assistenti sociali, cosa che avete rifiutato, e potenziando l'ispettorato del lavoro. Un tradimento, quindi, soprattutto verso le famiglie numerose e con persone disabili; un tradimento verso i bambini e le bambine che si attendono risposte coraggiose e durature nel tempo. Un tradimento verso i lavoratori precoci (parliamo di quota 100), verso le donne lavoratrici, verso i lavoratori con attività gravose e usuranti. Perché non avete indirizzato la vostra azione riformatrice verso quelle categorie maggiormente colpite dalla legge Fornero? Perché non farsi attenti verso coloro che nella propria vita non hanno potuto, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, avere una continuità contributiva? Le donne, per esempio, su cui spesso grava la cura nelle famiglie o le persone che hanno avuto prolungati problemi di salute. Avreste potuto fare tutto questo senza minare la tenuta finanziaria del nostro sistema contributivo, senza ipotecare il futuro delle migliaia di giovani che hanno il diritto di accedere a un trattamento pensionistico dignitoso.

dopo aver speso più di 20 miliardi di euro, tutti i problemi strutturali legati alla Fornero resteranno irrisolti, come pure quelli del *welfare* italiano. Avete introdotto a tempo un mero contributo e poco altro, perché alla fine questo provvedimento che a breve approveremo - che voi dite voi dite importantissimo, ci mancherebbe altro - si ridurrà a un mero trasferimento economico, molto piccolo, molto breve. La povertà non si sconfigge soltanto con trasferimenti economici - questa è una politica di destra; è stata sempre questa la politica di destra - ma si sconfigge nelle relazioni, nella presa in carico, non soltanto nel lavoro, in un piccolo sussidio economico, peraltro a tempo determinato. Le future generazioni saranno gravate da un debito pesantissimo:

vi aspettiamo tra qualche mese con la presentazione del Documento di economia e finanze, e poi con la prossima manovra. Ci spiegherete come questo provvedimento si sosterrà si sosterrà nei prossimi anni. Ahimè ci accorgeremo - spero di no soprattutto per le famiglie povere e per i pensionati più fragili e in difficoltà - che questo sarà stato un grande *bluff*, una grande promessa, un gioco

Finalmente verrà approvata quota 100 in via definitiva da parte del Parlamento alla sua seconda lettura: un punto fondamentale del programma della Lega; e verrà approvato il reddito di cittadinanza, punto fondamentale del programma del MoVimento 5 Stelle, nel pieno rispetto del contratto di Governo che ha portato alla formazione di questo Esecutivo. La prima questione che ritengo doveroso affrontare sono le critiche che sono state avanzate dalle opposizioni nei confronti di questo provvedimento: critiche mosse a quota 100 perché si doveva fare di più e si doveva fare meglio. Critiche prevedibili, ma - permettetemi - la domanda di fondo è un'altra: chi ha reso necessario un intervento legislativo per approvare questa riforma? Per essere più chiari, chi ha votato la legge Fornero? Non Certamente noi, non certamente la Lega. Proprio coloro che oggi criticano e giudicano il nostro operato, insegnano e danno lezioni. Permettetemi e perdonateci: lezioni da voi non ne possiamo accettare. I responsabili di quanto sta avvenendo in questa sede sono proprio le forze d'opposizione che oggi si oppongono nuovamente alla correzione e al superamento della legge Fornero. Avete avuto a disposizione cinque anni di Governo per rimediare agli errori commessi e alle ingiustizie che proprio voi avete approvato. Avete perso l'occasione e siete stati giustamente puniti dagli elettori. Nei vari dibattiti in quest'Aula e in quella della Camera avete criticato aspramente il reddito di cittadinanza affermando che è una misura sbagliata. La domanda però è sempre la stessa: dov'è la coerenza? Chi ha approvato poco più di un anno fa il reddito di inclusione e chi ha promesso in campagna elettorale l'approvazione di un reddito di dignità di 1.000 euro al mese, garantito per tutti? Le stesse forze politiche che oggi criticano un provvedimento che, anche grazie al contributo della Lega, non ha il solo obiettivo di aiutare le famiglie in grave stato di povertà, ma soprattutto l'obiettivo di far accedere al mondo del lavoro coloro che un lavoro lo hanno perso o non lo riescono ad ottenere. Il reddito di inclusione e di dignità delle opposizioni erano, quelli sì, puri provvedimenti assistenziali. Questo modello di reddito di cittadinanza investe sulla formazione, sui centri per l'impiego, prevede l'impegno a svolgere lavori socialmente utili, incentiva con la detassazione per le imprese l'assunzione di nuovo personale, prevede numerose prescrizioni affinché nessuno possa approfittare di questa opportunità. Non è, in definitiva, un provvedimento che elargisce denari a pioggia ma vuole essere uno strumento per dare slancio all'occupazione ed un futuro alle nuove generazioni. Sono state mosse poi altre critiche al provvedimento. L'Italia, è vero, si trova nuovamente in una condizione di crisi della crescita economica; è un dato reale e innegabile. È una situazione difficile per l'Italia e per l'Europa intera, Germania compresa. È stato più volte osservato che in questa situazione non era opportuno investire importanti risorse per la riforma del sistema pensionistico. Queste sono ovviamente le affermazioni delle opposizioni.

La modifica della legge Fornero è un atto di giustizia non più rinviabile ed è esattamente quello che noi oggi stiamo facendo in quest'Aula: un atto di giustizia. Stiamo restituendo una prospettiva di vita decorosa a uomini e donne cui è stata sottratta da una riforma profondamente ingiusta che proprio voi, tutti insieme, avete votato nel 2011. Il nostro percorso è totalmente diverso. La Lega, tutti noi senatori siamo coloro che non hanno dato la fiducia al Governo Monti. Siamo coloro che non hanno mai governato con il PD e con la sinistra; siamo coloro che hanno votato contro la legge Fornero; siamo coloro che hanno raccolto più di 500.000 firme per un *referendum* che cancellasse questa legge vergognosa. Siamo coloro che si sono battuti in Europa - lo voglio ricordare - perché quota 100 potesse trovare attuazione in una difficilissima legge di bilancio. Oggi, finalmente, ancora una volta in questa legislatura, siamo coloro che manterranno un impegno preso con i cittadini italiani. Noi non realizziamo questa riforma per la campagna elettorale delle elezioni europee: noi la realizziamo perché questo è il mandato che abbiamo ricevuto dagli elettori; un punto di partenza e non un punto di arrivo. Quota 100 è un atto di coerenza e di giustizia. È un atto di giustizia per i cittadini che hanno lavorato una vita intera e hanno il sacrosanto diritto di poter andare in pensione ad un'età dignitosa. È un atto di giustizia per dare il via ad un necessario ricambio generazionale nel mondo del lavoro mondo del lavoro e per ridare una speranza di vita ed un futuro in Italia ai nostri giovani. Avete insistentemente provato a difendere posizioni indifendibili, ma in definitiva voi dell'opposizione passerete alla storia per aver votato la legge Fornero nel 2011 e contro il suo superamento oggi. Siamo e potremo sempre dichiararci orgogliosi di non averla votata allora e di averla doverosamente smantellata oggi in quest'Aula. Ecco la verità dei fatti che rimarrà agli atti di questa legislatura e oggi finalmente giustizia è fatta.

avremmo desiderato e preferito che su questo provvedimento vi fosse stata un'apertura che avesse consentito a tutti i rappresentanti del popolo che siedono qui di portare il loro contributo.

Chi parla fa parte di un Gruppo parlamentare che ha dimostrato, nei fatti e non con le chiacchiere, non soltanto di essere sensibile ai problemi della povertà e del bisogno, ma anche di essere riuscito a risolverli.

e che non riguardano soltanto l'attività del Governo, ma i regolamenti, gli accordi con gli enti locali e quant'altro.

al cittadino di ritirare soltanto 100 euro al mese e vi preoccupate di stabilire come, quando e quali altri soldi dovranno essere spesi: questa è la democrazia partecipata che volete introdurre.

Ma la cosa clamorosa è che, per bocca del vice ministro Di Maio, il problema della povertà sarà risolto non soltanto con i soldi di tutti quanti (perché, ripeto,

evidenziare qualche differenza. In Germania vi sono 2.500 centri per l'impiego; in Italia ve ne sono soltanto 600. In Germania vi sono 110.000 addetti a tempo indeterminato con alto profilo culturale e professionale; in Italia ce ne sono 8.000,

cento dei contribuenti italiani dichiara un reddito inferiore a 10.000 euro annui, il 40 per Voi offrite 750 euro mensili a persone che non dovranno lavorare, sino a prova contraria, e andrete a mortificare centinaia di migliaia di lavoratori che mantengono le loro famiglie con una somma

di un popolo, quello meridionale, che si sente tradito dalle vostre promesse che sono state disattese e che quindi vi farà pagare un prezzo altissimo anche alle elezioni europee. Pertanto, quello che doveva essere il manifesto delle europee sarà un manifesto, sì, ma funebre del MoVimento 5 Stelle e della sua politica. Avete disposto cicli di audizioni, ma non avete ascoltato la parola, non dico delle opposizioni (in particolar modo di Forza Italia), ma neanche di quelle associazioni che hanno qualche titolo per parlare di di terzo settore e aiuto alla povertà. Non avete ascoltato la Comunità di Sant'Egidio, la Caritas e neanche Confindustria, che credo abbia qualche competenza nella creazione di posti di lavoro. Vi siete arroccati nelle vostre posizioni incomprensibili.

favolosa. Leggendo l'articolo 7-*ter,* che è stato introdotto alla Camera dei deputati, ci accorgiamo che il reddito di cittadinanza può essere dato anche ai pregiudicati e ai latitanti,

Ma vi è di più! Un partito che ha fatto dello "spazza corrotti" un cavallo di battaglia si trova nella

non è una contraddizione, è un filo logico. Il MoVimento 5 Stelle vuole fuori dalle amministrazioni della politica i corrotti; però, siccome anche i corrotti tengono famiglia, vuole dare loro il reddito di cittadinanza, a carico di tutti gli italiani! Complimenti! Presidente, due parole anche su quota 100. Amici della Lega, diciamo le cose come stanno. Questa quota 100 non supera affatto la legge Fornero e, probabilmente, fra tre anni l'avremo nuovamente, aggravata dei debiti che state creando. Infatti, un *record* l'avete raggiunto: aumentate di sei miliardi al mese il debito pubblico. Questo è il vostro primato! La quota 100 è soltanto un beneficio temporaneo, che si applicherà per tre anni a pochi fortunati e che

c'era la misura del superammortamento del 130 Dov'è andato a finire il 130 per cento di superammortamento? Valutando in 30 miliardi la spesa per quota 100, se fosse stata impiegata per il superammortamento al 130 per cento, e valutando un contributo

Allora, agli amici della Lega dico: "chi troppo in alto sal, sovente cade". Meditate, colleghi della Lega. Noi ve lo abbiamo detto. Non potete dire che non ve l'abbiamo detto. E, per darvi un contributo di resipiscenza, voteremo in maniera convinta no a questo provvedimento!

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, 1.974 giorni: tanti ne sono passati da quando, il 29 ottobre 2013, abbiamo presentato, proprio qui in Senato, il primo disegno di legge per l'istituzione del reddito di cittadinanza, a prima firma della senatrice Nunzia Perciò, signor Presidente, colleghi, oggi è un giorno storico: per il MoVimento 5 Stelle, per chi l'ha fondato, per chi, in questi anni, ha portato avanti, con coraggio, tante battaglie, ma soprattutto per l'Italia intera. Oggi, infatti, milioni di cittadini che, giorno dopo giorno, sono stati dimenticati, lasciati volutamente (ribadisco, volutamente) ai margini da una politica cieca e sorda agli epocali cambiamenti avvenuti, senza prendere le adeguate contromisure, sanno che possono contare sullo Stato. Uno Stato forte, che tende loro la mano, invitandoli a stringere un nuovo patto sociale, restituendo loro la dignità perduta e ridando loro la speranza nel futuro. Lo dico senza troppi giri di parole. Vista la cruciale portata di questo provvedimento, ci saremmo aspettati che oggi l'Assemblea del Senato lo votasse all'unanimità, soprattutto la sinistra che invece, in maniera sprezzante, ad un certo punto, con qualche illustre esponente, ha persino ironizzato, parlando dei futuri beneficiari del reddito di cittadinanza come di poveri che avrebbero passato la loro vita in vacanza. Addirittura c'è chi ha lanciato l'idea di raccogliere le firme per un *referendum* contro il reddito di cittadinanza, cosa che peraltro, in una riedizione del famigerato patto del Nazareno, ha detto di voler fare anche la destra. Siamo proprio curiosi di sentire cosa direbbero se si trovassero di fronte Salvatore che a sessantadue anni, dopo una vita di lavoro come muratore, tre anni fa si è ritrovato improvvisamente senza più niente e oggi, purtroppo, vive chiedendo l'elemosina e mangiando alla Caritas; o se dovessero incontrare Francesco, che a ventidue anni è stato costretto a mettere in secondo piano gli studi per un lavoro saltuario che non lo facesse pesare sui suoi genitori; o ancora davanti a Cesare che a cinquantadue anni, dopo la chiusura dell'azienda nella quale era impiegato, fa le pulizie per meno di 250 euro al mese con i quali deve dare da mangiare a sua moglie e a suo figlio; per non parlare di Matteo che prende 450 euro al mese di pensione e ha un figlio disoccupato. Non solo sono storie vere queste. Questi, signori, sono solo alcuni esempi del Paese che ci hanno lasciato i vecchi Governi, un Paese passato da due a oltre cinque milioni di persone in povertà assoluta, proprio negli anni in cui questi stessi Governi andavano in Europa con il cappello in mano, facendosi imporre delle politiche economiche da macelleria sociale. *(Applausi anni in cui abbiamo sentito Ministri dare dei bamboccioni e degli sfigati ai nostri ragazzi, dicendo che per loro, per poter trovare lavoro, era era meglio giocare a calcetto che mandare *curriculum*. Ma vi rendete conto? Noi oggi, con questa riforma che tra i punti qualificanti ha un investimento senza eguali in politiche attive del lavoro, diciamo a questi stessi ragazzi: andate nei centri per l'impiego, perché finalmente non rappresenteranno più un'umiliazione per voi e per quelle tante persone che in questi anni si sono rivolte ad essi, mescolando rabbia a frustrazione. mentre i vecchi Governi investivano lo 0,05 per cento del PIL in servizi per il lavoro, Francia e Germania mettevano sul piatto rispettivamente cinque e sette volte più di noi. E meno male che siete quelli competenti. Fortunatamente quel tempo è finito. Una volta al Governo, il MoVimento 5 Stelle ha messo al centro della propria azione politica i cittadini e i loro reali bisogni, un'azione che ha avuto come direttrice e fondamento la tutela e la garanzia della dignità di tutti i cittadini i quali hanno pari dignità sociale, come è scritto nell'*incipit* dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Per troppo tempo questo assunto è stato dimenticato, sacrificato sull'altare del profitto e della globalizzazione sfrenata. Molti di voi, cari colleghi, si sono abituati alla brutale idea che chi è povero deve restare e morire povero ma non noi che infatti, come primo provvedimento, una volta arrivati al Governo abbiamo varato proprio il cosiddetto quello che a detta dei detrattori avrebbe provocato l'apocalisse e invece gli ultimi dati ci dicono che c'è stato un vero e proprio *boom* di trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Adesso, questo percorso continua con il reddito di cittadinanza che ha come Stella Polare quella parola, carica di significato e di responsabilità per chi amministra il Paese, che è presente sempre nella nostra Costituzione, stavolta all'articolo 1: lavoro. Anche su questo punto la vostra fantasia si è scatenata: pur di non voler ammettere che con questo provvedimento chi oggi si ritrova fuori dal mercato del lavoro potrà godere di una nuova opportunità, frutto di un serio percorso di formazione e riqualificazione, ne avete dette di La verità invece è che nessun Governo prima del nostro aveva mai investito così tanto in servizi per il lavoro per colmare quel *gap* che ci separa dai principali *partner* europei. Con questa riforma cominciamo a portare in Italia il livello di Germania e Francia, nei cui centri per l'impiego lavorano rispettivamente 100.000 e 54.000 addetti. Addirittura negli uffici locali tedeschi operano i consulenti per il lavoro, 6.000 dei quali specializzati nei rapporti con le imprese: numeri incredibili se confrontati con quelli del nostro Paese, che solo grazie a questo intervento, dopo anni di immobilismo, vedrà aumentare significativamente il numero dei propri addetti che al momento sono solo 8.000. L'investimento non sarà solo in capitale umano, ma anche in infrastrutture tecnologiche per mettere finalmente in comunicazione domanda e offerta di lavoro. Se questo processo fosse iniziato anni fa, se ci aveste dato ascolto quando da questi banchi gridavamo l'urgenza di istituire il reddito di cittadinanza, oggi oggi saremmo sicuramente un passo avanti. Ma come si dice: meglio tardi che mai. Con questa misura, come diceva qualcuno a noi molto caro, nessuno resterà più indietro. Solo così possiamo ricostruire quel senso di comunità che questo Paese ha perduto. Solo così possiamo riattivare il motore della crescita, un possiamo riattivare il motore della crescita, un motore grazie al quale guideremo l'Italia verso un futuro fatto di diritti e opportunità. Crescita e futuro: sono i due pilastri del provvedimento in discussione e della futura azione di Governo con la fissazione del salario minimo orario. Infatti, è possibile rilanciare la produttività e i consumi solo emancipando i cittadini dalla condizione di bisogno. Il combinato disposto di reddito di cittadinanza e salario minimo orario avrà effetti positivi sull'economia, in quanto aumenta il potere d'acquisto per i lavoratori, rilancerà i consumi e conseguentemente alimenterà la domanda interna, con più profitti per le imprese, alle quali saranno destinate ulteriori misure di riduzione del cuneo fiscale. Con questo provvedimento mandiamo in porto anche un altro dei punti qualificanti del nostro programma e del contratto di Governo, ovvero quota 100. La legge Fornero ci è costata carissima, sia in termini sociali che economici. Vedere per credere quanto lo Stato ha speso per le varie salvaguardie. Nei prossimi tre anni un milione di lavoratori avrà la possibilità di andare in pensione anticipatamente, aprendo al ricambio generazionale, tanto nel pubblico impiego quanto nel settore privato. Abbiamo confermato APE sociale e opzione donna, altre due misure importanti. Signor Presidente, tornando al reddito di cittadinanza desidero citare i nostri fondatori, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. *(Applausi Il primo ha sempre detto che «il reddito di cittadinanza è vedere il mondo del lavoro in un altro modo, è un diritto civile»: si tratta di dare un'occasione alla gente. Il secondo sosteneva «togliere dalla disperazione e dalla povertà milioni di poveri è un obbligo morale», «una battaglia di civiltà in cui le appartenenze politiche devono scomparire». Con queste frasi, che sono state la nostra guida nel percorso di genesi e realizzazione del reddito di cittadinanza, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

il Governo non ha ancora compensato i danni subiti da tante famiglie e imprese veronesi a causa dell'alluvione dello scorso 1° e 2 settembre. Il 27 febbraio scorso è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce le risorse per fronteggiare i gravi eventi calamitosi che si sono verificati in diversi Comuni del Paese; quindi la realizzazione di investimenti strutturali e infrastrutturali per compensare i danni che quegli eventi hanno provocato. I beneficiari delle risorse nel Paese sono i territori colpiti da eventi atmosferici eccezionali accaduti negli anni 2017 e 2018. Il decreto però esclude i Comuni di Verona, Negrar, San Pietro in Cariano, Colognola ai Colli, San Martino Buon Albergo, Zevio, Belfiore, Soave, Monteforte d'Alpone, Cazzano di Tramigna e Illasi, ovvero Comuni che sono stati colpiti da una grave alluvione nei giorni 1° e 2 settembre 2018, per i quali peraltro la Regione Veneto aveva già dichiarato lo stato di crisi e richiesto lo stato di emergenza, lo stato di emergenza, decretato dal Consiglio dei Ministri il 17 gennaio scorso. Perché il Governo ha escluso Verona? Sono in corso le procedure per stanziamenti mirati?

Presidente, voglio qui segnalare il fatto, sollecitando l'urgente necessità di riesaminare la posizione del Governo, ovvero il diniego finora ricevuto, al fine di non discriminare il territorio veronese interessato da questi eventi rispetto ad analoghi accadimenti avvenuti

il mio intervento è volto a segnalare a quest'Assemblea e al Governo la situazione di criticità e le problematiche relative alla circolazione dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci sulla *route départementale* 6204 della Val Roia, che si collega, nel tratto italiano, alla strada statale 20 del Colle di Tenda, che interessa il trasporto e lo scambio di merci tra le Regioni Piemonte e Liguria e il Sud-Est della Francia.

presentarono presso la prefettura di Nizza un'ordinanza congiunta, con la quale decretarono la limitazione sulla strada 6204 nei rispettivi territori municipali ai veicoli aventi massa massima superiore alle 19 tonnellate. Un'ordinanza generica, che indica in modo assolutamente scorretto ai trasportatori di scegliere quali itinerari alternativi - udite bene - il tragitto sulle autostrade A6 e A10, con un aggravio di sette ore in più per viaggio e di 180 euro di costo in più per viaggio e con un allungamento del viaggio per i mezzi pesanti di ben 200 chilometri. È scritto sul divieto che tempi e tragitti alternativi sarebbero minimi. Queste assurde considerazioni, messe nero su bianco nelle ordinanze, non sono state supportate da alcun dato statistico sul reale utilizzo di questo valico strategico per il nostro Paese, ma anche per la Francia. Le cinque municipalità francesi interessate di fatto collocate in una lingua di territorio in cui transita una via di comunicazione internazionale, non una stradina comunale; è una via di importanza vitale. Considerata la gravità del provvedimento emanato dai sindaci della Valle Roia, ritenuto da noi inopportuno e in contrasto con gli interessi produttivi e commerciali delle Regioni interessate, noi ribadiamo la richiesta di ritiro e di annullamento dell'ordinanza, come già espresso dalle associazioni di categoria e dalle imprese produttive italiane. Le stesse imprese che il 18 marzo, in occasione della visita del presidente Conte e del ministro Toninelli in quel di Cuneo, hanno sollecitato questo provvedimento;

iscritto a parlare il senatore Aimi. Signor Presidente, lo scorso 10 marzo in Sardegna, sulla strada provinciale che collega il centro abitato di Siniscola alla vicina frazione Marina della Caletta, ha perso la vita Emanuele Tancale, un ragazzo di diciotto anni, travolto da un'auto mentre con un amico rientrava a casa a piedi dopo aver partecipato ai festeggiamenti del carnevale. Alla guida dell'auto c'era un altro ragazzo come lui, di ventidue La tragedia è avvenuta su una strada provinciale; una strada come tante in Italia, una di quelle strade che portano verso il mare, che d'estate i ragazzi percorrono con gli *scooter*, in bicicletta o a piedi. È una strada pericolosa, come tante altre strade provinciali in Italia: un rettilineo di 5 chilometri senza illuminazione, dove si affacciano ingressi di abitazioni private, una scuola, dove convergono altre strade, con scarsa segnaletica orizzontale e verticale, senza marciapiedi, con una carreggiata troppo stretta, soprattutto per l'ingente afflusso e traffico estivo. Una strada provinciale in stato di abbandono, come tante in Italia, a causa dei tagli delle risorse subiti negli ultimi anni dalle Province, realizzati nel tentativo di soffocare gli enti territoriali cosiddetti di Area Vasta. Oggi, signor Presidente, voglio esprimere la mia vicinanza, da siniscolese, alla famiglia di Emanuele Tancale, alla madre Antonella, al padre Gianfranco; voglio esprimere la mia vicinanza anche a Maria Antonietta, la madre del ragazzo alla guida dell'auto, tutti, seppur in modo diverso e da diversi punti di vista, vittime di un dramma. Ma vorrei anche invitare tutti ad una riflessione. La nostra attenzione, l'attenzione dei *media*, ultimamente è stata catalizzata dai dubbi sull'opportunità di realizzare alcune grandi opere. Credo sia necessario pensare nuovamente e con maggiore attenzione anche alle piccole opere, piccole opere, fondamentali per la sicurezza nostra e dei nostri cari. Quante sono le strade provinciali che percorriamo durante l'anno? Quante sono le strade provinciali che percorrono i nostri amici, i nostri familiari, i nostri figli,

Signor Presidente, cari colleghi, sottopongo oggi alla nostra attenzione e all'attenzione dell'Assemblea un tema che sta a cuore ai cittadini, al di là delle bandiere politiche. Parliamo di sanità, quindi di diritto alla salute. In Veneto, in provincia di Padova, la casa di cura di Abano rischia di essere declassata da ospedale a struttura integrativa della rete ospedaliera pubblica. In parole povere, ciò comporta comporta una riduzione di servizi, quindi una penalizzazione per i nostri cittadini. Vuol dire riduzione del numero delle prestazioni erogate, sia sia ai cittadini residenti, sia a tutti i visitatori di un'area turistica come quella delle Terme euganee, con più di 3 milioni di visite all'anno. Vuol dire chiudere il pronto soccorso, che ogni anno registra 38.000 accessi. Rischiano di chiudere anche la terapia intensiva, la traumatologia, l'ostetricia, la rianimazione e tutta una serie di altri servizi. Parliamo di numeri, ma anche di qualità, e soprattutto di persone. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenas, l'ospedale di Abano è tra i primi in Italia come qualità dell'assistenza nell'ambito della chirurgia della prostata e della chirurgia del ginocchio. È impensabile che le centinaia di migliaia di turisti (circa 800.000 ogni anno) che visitano il bacino euganeo debbano far riferimento per i servizi di urgenza e pronto soccorso a strutture ospedaliere, come l'ospedale di Schiavonia o quello di Padova, raggiungibili nelle ore di punta dopo più di un'ora. Non si toccano i servizi ai cittadini. Come si può pensare di chiudere una struttura che registra 42.000 utenti all'anno? Alla Presidenza e a tutti voi, colleghi, intendo porre questa situazione che - ne sono certo - è solo un esempio di disinvestimento rispetto al nostro sistema sanitario, che necessita di un piano di di intervento strategico, possiamo dire di un "piano Marshall". Mi avvio alla conclusione, ponendo all'attenzione di quest'Assemblea il tema della *spending review* in sanità. Bisogna cambiare rotta: non è possibile disinvestire sul diritto alla salute; bisogna tornare a investire sulla salute dei nostri cittadini. Credo che questo sia un tema da cui non possiamo prescindere, come dicevo all'inizio, indipendentemente dai colori e dalle appartenenze politiche. Lo faccio perché, come è noto, a livello nazionale ormai da anni si registra una pesante carenza di medici, infermieri e personale sanitario, sia nei nostri ospedali al Nord Grazie che in tutto il mondo, nonostante le criticità e le differenze a livello territoriale, ci invidiano. Stipulare dei contratti ai medici in pensione, come sta avvenendo in questi giorni in alcune Regioni, è sicuramente una soluzione, ma è solo una soluzione tampone.

lo dicono i numeri. Secondo l'Anaao Assomed, in Italia nei prossimi cinque anni mancheranno 45.000 medici. Sempre secondo le associazioni, stando ai recenti dati dell'Eurostat, negli ospedali italiani nel 2016 operavano circa 213 medici ogni 100.000 abitanti, cifra che sale in Francia a 264, in Germania a 237, in Spagna a 227 Ma la situazione nazionale rischia di passare a 181 medici ogni 100.000 abitanti entro il 2025: una situazione che non può reggere per la sanità e per la salute dei nostri cittadini. Bisogna quindi rivedere il sistema di formazione dei medici nelle nostre università e il numero chiuso. Occorre investire più risorse nelle scuole di specializzazione e serve anche un nuovo modello nel servizio sociosanitario; serve più personale parasanitario. Oggi i medici passano troppo tempo a occuparsi di burocrazia. C'è un problema di risorse e investimenti. Disinvestire sul diritto alla salute è una scelta sbagliata. *(Applausi Grazie l'associazione "Italiadecide - Associazione di ricerca per la qualità delle politiche pubbliche", presidente Luciano Violante, qualche giorno fa ha premiato alla Camera dei deputati, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella, la società per azioni Abbanoa, il cui capitale è interamente pubblico, la quale gestisce *in house* l'intero servizio idrico integrato sardo. «Un efficace esempio di recupero di una situazione deficitaria scarsamente industriale e frammentata che ora marcia su un profilo di efficace e sana gestione»: con queste motivazioni ad Abbanoa è stata riconosciuta la menzione speciale per il prestigioso Premio Italiadecide, riservato quest'anno alle società pubbliche dei servizi idrici integrati. È vero che Abbanoa ha consentito di superare il servizio gestito da amministrazioni comunali e società deficitarie e in liquidazione, ma la riorganizzazione e il risanamento societario, come l'ammodernamento delle strutture, lo hanno pagato amaramente i cittadini sardi, e non soltanto i termini di più elevati costi, ma anche di disservizi gravissimi. Sono anni che i cittadini sardi combattono, persino nelle aule dei tribunali, contro fatture assurde, con importi davvero da infarto per costi di servizi mai erogati conguagli pregressi, contro minacce e talvolta lo slaccio a intere famiglie impossibilitate a pagare queste esose, talvolta ingiustificate, fatture. Interi condomini lasciati senza acqua per la morosità di alcuni condomini, acqua non potabile, gialla o *marron*, che sgorga per giorni dai rubinetti di intere città a causa delle condotte ormai vetuste, non parlare di quando interi paesi sono stati lasciati per giorni completamente senza acqua, persino durante la stagione estiva. Abbanoa ha perso diverse cause davanti ai giudici, che l'hanno condannata a risarcire ai cittadini i danni da essa arrecati la stessa *Antitrust* le ha inflitto una sanzione di 680 milioni di euro per pratiche aggressive e vessatorie nei confronti dei cittadini. Ciò detto, conferire ad Abbanoa un premio per sana ed efficiente gestione appare davvero una barzelletta agli occhi di tutti i sardi. Sembra un'operazione sostenuta da una certa area politica, che ha bisogno di gratificarsi da sola per biechi fini propagandistici.

Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, ieri è stato un giorno nero per la libertà in Internet, a causa dell'approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva sul *copyright*, contro cui in questo fine settimana hanno manifestato decine di migliaia di persone ed è stata firmata una petizione con milioni di firme. Anche "Wikipedia" ha oscurato le proprie pagine per dare visibilità alla protesta. C'è chi ha detto che il 26 marzo 2019 il *web*, per come lo abbiamo conosciuto, è morto: creato nel 1989 da uno scienziato, Tim Berners Lee, e distrutto dopo trent'anni, nel 2019, da un politico, Axel Voss, relatore di questa pessima riforma. Una delle migliori invenzioni dell'uomo è stata mutilata dalla politica, probabilmente per mancanza di conoscenze tecniche o per semplice ignoranza. Per una persona come la sottoscritta che ha partecipato attivamente alla nascita e alla realizzazione di Internet in Italia, questa direttiva dimostra come, fino all'ultimo, l'attuale classe politica europea che ancora per poche settimane avremo a Bruxelles e a Strasburgo - invece di tutelare i diritti e le libertà dei cittadini preferisca in realtà schierarsi a favore della *lobby* degli editori. Il *web,* fin dalla sua nascita, ha rappresentato una rinata opportunità per tutti di collocare il diritto di scrittura sullo stesso piano del diritto di lettura, il diritto di produrre informazione sullo stesso livello di quello di ricevere informazione. Il *web* è la possibilità tecnico-economica di esercitare questi diritti. Questa direttiva tende invece all'introduzione per legge dell'asimmetria: solo pochi hanno il diritto di informare, mentre tutti hanno il diritto di ricevere informazioni, da pochi *content provider*. I pochi che mantengono il diritto di informare sono coloro per i quali sarà conveniente pagarne i diritti d'autore. Oltre ai dubbi sulle difficoltà di recepimento, dovuti ai lunghi tempi tecnici, che non permettono di sapere se tali regole saranno ancora utili in futuro e alla vaghezza e approssimazione di alcune norme, che avranno come conseguenza leggi diverse per ogni Stato membro dell'Unione europea, l'aspetto più grave è che non esiste un solo studio di impatto della nuova disciplina sul mercato editoriale e su quello dei contenuti creativi *online*. Il rischio concreto è che la riforma trasformi i gestori delle grandi piattaforme, che sin qui hanno ospitato contenuti prodotti dagli utenti, in editori. La mia speranza e quella di tanti altri, che condividono la mia visione, è che l'attuale Governo che si era espresso contro la riforma, definisca al meglio i contorni esatti di questa nuova riforma, in modo che vengano esaltati i pochi aspetti positivi e limitati quelli fortemente negativi, al fine di tutelare i veri sconfitti di ieri, che non sono i giganti del *web*, ma i cittadini europei, i quali hanno un'ultima possibilità: cambiare la classe politica alle prossime elezioni europee.